mozioni sulle riforme costituzionali predisposte e presentate da tutti i Gruppi del Senato

Da molti decenni ormai la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (cioè il Parlamento italiano) hanno avviato, con le modalità più varie, processi di riforma della Costituzione. È largamente prevalente nel Paese e nel Parlamento l'idea che la Costituzione della Repubblica italiana, a sessant'anni dalla sua promulgazione, sia tuttora moderna e funzionale, ma è altrettanto diffusa nel Parlamento l'idea che, soprattutto nella seconda parte della Costituzione, siano necessari aggiustamenti, modifiche e riforme che, nel mantenerne lo spirito, rilancino in qualche misura l'efficacia e l'efficienza del sistema democratico in una società che si è profondamente modificata nel corso degli anni. Per questa ragione, e nella considerazione che nel corso di questi decenni i tentativi posti in essere, anche con spirito assai costruttivo (desidero ricordarne due in particolare: la Commissione Bozzi e la Bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema), arrivarono a risultati molto avanzati anche in termini di consenso e poi, per incidenti politici vari, non riuscirono ad arrivare al risultato,

2). Lo scopo fondamentale della nostra mozione e del dibattito che oggi si avvia, signor Presidente, è non pensare che rispetto alle necessità di adeguamento della Costituzione si possa procedere

costituzionali, assecondando una modifica radicale della Costituzione materiale, che non è stata mai approvata da nessuno dei due rami del Parlamento, ma che di fatto ne stravolge le regole fondamentali.

fatto che le modifiche alla Carta costituzionale, cioè la riforma della Costituzione, non possono che essere scritte da una larga maggioranza. Nel corso degli ultimi dieci anni, con modalità assai diverse, in Parlamento si è proceduto all'adozione di modifiche della Costituzione

Nella successiva legislatura, la maggioranza di centrodestra di allora, l'attuale maggioranza, arrivò ad una riscrittura totale della Costituzione, sostanzialmente da essa sola condivisa. Oggi il punto politicamente di maggiore rilievo politicamente di maggiore rilievo è che tutte le mozioni riconoscono che a tale processo di revisione della Costituzione occorrerà lavorare tutti insieme, a partire - come diciamo nella nostra mozione - dalla necessità di mettere mano a quelle modifiche che la Camera dei deputati approvò nella scorsa legislatura con l'Atto Camera 553 e proposte abbinate (la cosiddetta bozza Violante), che dovrebbero interessare anzitutto la riduzione del numero dei parlamentari per riportarlo su un media compatibile con quella delle altre grandi democrazie, ma anche condurre alla modifica e al superamento del bicameralismo perfetto, del bicameralismo paritario, con la trasformazione del Senato nel Senato federale della Repubblica. Presidente, questo non vuol dire evidentemente che i senatori del Partito Democratico - e mi avvio a concludere - scelgano il modello adottato da quella Camera nella scorsa legislatura. Avvertiamo l'esigenza di approfondire con grande serietà le modalità attraverso cui il Senato possa diventare sempre più un Senato specializzato in una funzione normativa in rapporto con il territorio; le modalità attraverso cui tale compito deve essere espletato ovviamente saranno oggetto di valutazione. Né pretendiamo, Presidente, che l'elenco sia esaustivo: mancano alcune questioni di grande rilievo. Ne voglio citare una per tutte: quella della legge elettorale.

Oggi la mancanza di forza, di autorevolezza e di prestigio del Parlamento deriva anzitutto da una legge elettorale che in qualche misura lo delegittima. Rispetto a tutto questo credo si possa dire che oggi la ripresa., l'avvio di tale dibattito sia un momento importante della vita di questa legislatura. *(Applausi

pochi minuti per illustrare una mozione dal contenuto essenziale e stringato, opportuno in questi termini perché, se si vuole aprire un dibattito, così come fa anche in modo analogo la mozione del PD, occorre che i temi vengano individuati, ma che siano necessariamente sfumati. Tuttavia alcune premesse vanno fatte. Innanzi Innanzi tutto, e questa credo sia una valutazione condivisa, il nostro sistema costituzionale è alla ricerca di nuovi equilibri,

ad altri livelli ed anche a livello della società civile. Gli equilibri costituzionali sono condizione necessaria, anche se non sufficiente, per una convivenza civile regolata e per uno sviluppo ordinato. Certamente, lo squilibrio si è accentuato alla fine degli anni '80 e al principio degli anni '90, con la

Certamente, questa Costituzione non è quella del 1948. Essa ha subito modifiche importanti e rilevanti, alcune condivisibili ed altre no, alcune efficaci ed altre problematiche.

abbiamo i governatori, abbiamo un sistema di autonomie molto significativo. A fronte di Governi regionali molto forti, però, abbiamo un Governo nazionale molto debole. Quindi, occorre riequilibrare anche nel sistema complessivo la presenza del Parlamento e l'espressione, da parte del Parlamento,

principio della sussidiarietà del quale il federalismo è un'espressione, ma ha anche creato - riconosciamolo - una grande confusione di ruoli e una grande conflittualità, che danneggia soprattutto gli enti

non ha più ragione di esistere. Credo che questa Camera ci debba essere e debba avere la dignità di una Camera rappresentativa di livello nazionale e di organo di raccordo e di mediazione tra lo Stato e le autonomie.

Presidente, onorevoli colleghi, parto da un rilievo formale,

Utilizzare però la formula dell'impegno al Governo per proporre una discussione su un tema costituzionale mi appare francamente come una sorta di spoliazione volontaria propria potestà da parte del Parlamento e una sorta di interlocuzione con un soggetto che in realtà, in questo caso, dovrebbe essere a lato, se non addirittura assente. La discussione sulla riforma costituzionale è potestà dell'Assemblea parlamentare, delle Assemblee elettive, e non c'è alcun bisogno dell'interlocuzione con il Governo, né c'è bisogno dell'autorizzazione del Governo per discutere di una cosa simile. simile. L'evidenza della potestà della discussione parlamentare su temi costituzionali

l'appoggio del popolo, in proporzioni indiscutibili, alla Carta costituzionale così com'era stata scritta dai Padri costituenti. Essa non era stata approvata all'origine, perché non ce n'era stato bisogno. Dopo qualche generazione, gli italiani hanno potuto prendere cognizione della Carta

Questo voto ha un valore fondativo, un valore originario: esso rimette in primo piano la Costituzione così com'era e la sottrae alla contingenza di una discussione politica che vuole immaginare la sua trasformazione sulla base di necessità, queste sì, veramente limitate, occasionali e contingenti. Se si deve discutere di riforma della Costituzione, non ci si può basare su termini così episodici, limitati e frammentari come - così si dice - il conflitto tra politica e giustizia. Il tema del conflitto tra politica e giustizia è del tutto estraneo al dibattito intimo sulla questione costituzionale. Si può discutere di riforma della Costituzione perché, nonostante e sulla base del voto del 2006, si ritiene che debbano essere apportati degli aggiustamenti minimi, che non devono ledere in nessun caso il quadro complessivo delle garanzie, che non devono ledere in nessun caso il quadro degli equilibri costituzionali tra i poteri costituzionali, che non devono rimettere in discussione nulla del sistema complessivo, fondativo della Costituzione. Si può discutere di aggiustamenti della Costituzione dal punto di vista della funzionalità di certi aspetti dell'ossatura istituzionale della situazione italiana, ma non si può partire dalla occasionalità di fattori di polemica e di conflitto politico per indurre che solo con l'ingegneria costituzionale si possono risolvere i problemi politici. È questo il tema fondamentale, il discrimine tra una visione pura dell'argomento e una visione opaca.

Ma il quadro delle garanzie costituzionali, il quadro dell'equilibrio tra i poteri costituzionali deve essere lasciato esattamente intatto, così come il voto popolare l'ha riconfermato e in un certo senso ricostituito. Tutti i diritti che nella vita quotidiana si avvertono come fondamentali devono essere risolti nel quadro dei diritti costituzionali, ma non ricevono una risposta diretta dalla Costituzione, né dalla riforma costituzionale. Il lavoro, l'istruzione, il diritto l'autodeterminazione, la capacità di scelta, la parità delle opportunità, la difesa dell'ambiente, il rilancio dell'economia: non si può dire che c'è bisogno di una riforma istituzionale per cambiare. Bisogna puntare ad una riforma costituzionale che aggiusti ciò che vi è da aggiustare. Cosa c'è da aggiustare? Ben poco, veramente ben poco. si possa immaginare una riduzione del numero dei parlamentari, costruire un Senato diverso da quello che la Carta costituzionale aveva disegnato, ma non si può pensare di passare attraverso questo trucco per sostenere che bisogna rafforzare il potere dell'Esecutivo. Se c'è una cosa di cui in Italia non c'è assolutamente bisogno è rafforzare il potere dell'Esecutivo e poiché tra

Noi pensiamo, ad esempio, che si possa avere un atteggiamento riformistico su aspetti di cui ogni tanto si viene accusati. Siamo individuati dall'opinione pubblica come il partito delle manette: non sto a smentire tale affermazione, ma nella nostra idea di riforma costituzionale immaginiamo, ad esempio, che si possa stabilire che i magistrati che sono entrati in politica

I *referendum* abrogativi possono essere modificati in maniera molto semplice: aumentando il numero dei richiedenti e, nello stesso tempo, sopprimendo l'idea del *quorum*. In fondo, molti *referendum* su argomenti seri sono stati letteralmente ammazzati dal fatto che forze politiche interessate a farli fallire hanno determinato semplicemente un'astensione preventiva che ha reso vana la consultazione.

e poniamo ciascun elettore di fronte alla necessità di pronunciarsi: chi vuole veramente decidere va a votare, chi non vuole decidere non si reca a votare, ma non diventa però neppure il soggetto che, non decidendo, impedisce agli altri di decidere.

ledendo, smantellando ed incidendo sul rapporto tra i poteri costituzionali. In conclusione - lo ripeto, perché fa parte della nostra convinzione più radicata non accetteremo mai alcuna procedura che porti ad un rafforzamento dell'Esecutivo, neppure in quella forma surrettizia per cui si dice, di solito: rafforziamo l'Esecutivo e rafforziamo i poteri del Parlamento.

del Parlamento. Nella situazione italiana, però, viziata da un'anomalia istituzionale senza precedenti in nessun Paese democratico, non è lecito liberare l'immaginazione fino a questo punto: il rafforzamento dell'Esecutivo rappresenta per forza una conculcazione della potestà delle Assemblee elettive. Quindi, se un potere deve prevalere, è quello del Parlamento e non certo quello di un Governo che, come tale, è sempre transeunte.

ha stilato una Costituzione caratterizzata da una grande anima sociale e democratica, in cui suggella i diritti e le libertà fondamentali, che la distinguono tra le più avanzate delle democrazie moderne. L'ordinamento organizzativo, invece, seguiva una chiara traccia centralistica: era sì prevista la presenza delle Regioni, ma senza che fossero loro attribuite competenze esclusive proprie. I Padri temevano una frammentazione in tanti piccoli staterelli, frammentazione dalla quale, con l'unificazione d'Italia, si era finalmente usciti. Le uniche eccezioni in questo sistema furono le Regioni a statuto speciale, costituite per affrontare le particolarità e i problemi che si presentavano nei loro territori per motivi storici, politici e culturali. A partire dagli anni '80 sono stati intrapresi vari tentativi per una riorganizzazione dello Stato. Gli inizi risalgono al 1983, alla cosiddetta Commissione Bozzi. Negli anni '90 la spinta propulsiva proveniva dalle Regioni, che avevano sviluppato una maggiore consapevolezza della propria identità, e dall'allora nuova forza politica, la Lega Nord, che chiedeva una riforma dello Stato in senso federale. furono i tentativi falliti: ricordo le Commissioni e le proposte Labriola nel 1991, De Mita e Iotti nel 1992 e quella D'Alema, pure vittima di una crisi di Governo, però ripresa dallo stesso, quale Presidente del Consiglio dei ministri, che, nel 2001, portò finalmente ad una riforma. riforma del 2001 va a toccare il nucleo dell'ordinamento statale e cioè gli enti che formano la Repubblica, escludendo però - e lo sappiamo tutti - vari aspetti importanti che dovrebbero far parte di una vera riforma in senso federale. Le Camere sono rimaste immutate, senza che sia stata prevista una Camera delle Regioni. Condividiamo pertanto in linea generale i principi elencati nelle mozioni qui presentate. Sottolineo positivamente soprattutto i seguenti aspetti: che la riforma costituzionale avvenga con spirito leale di collaborazione nel confronto parlamentare e con che venga ridotto il numero dei parlamentari, che permette di abbassare non solo i costi della politica e dell'apparato burocratico, ma anche di semplificare il dibattito parlamentare. Come terzo punto mi pare importante riservare una delle due Camere previste nel nostro ordinamento alla espressione democratica delle istanze regionali, completando un ulteriore tassello che qualifica un vero Stato federale Su questo punto vorrei porre però un forte distinguo nel peso istituzionale e politico che si dovrebbe attribuire a questa seconda Camera. Al riguardo, vorrei che i senatori presenti in questa Camera si rendessero conto della domanda che ci poniamo. Il progetto Il progetto espresso di superare il cosiddetto bicameralismo perfetto si riferisce ad esperienze della vicina Austria e della Germania, in cui le Camere hanno competenze diverse, senza però tener conto delle critiche e delle debolezze di questi sistemi, che stanno facendo riflettere i costituzionalisti di quei Paesi. In un seminario che ho avuto l'onore di tenere all'università di Vienna sullo sviluppo del federalismo in Italia, nella discussione mi è stata posta la seguente domanda, anche per me allora sorprendente. Mi si chiedeva: per quanto sia apprezzabile che l'Italia, con grande ritardo, si appresti a creare una Camera di espressione federale, avete tenuto conto delle critiche che sono maturate nei Paesi che questo sistema lo applicano da decenni? critiche nei Paesi dove c'è questa seconda Camera. Non avrete mica l'intenzione - questa era la domanda centrale - di compiere lo stesso errore che è stato compiuto in Austria ed anche in Germania, di creare cioè una Camera senza reali che di fatto influisce pochissimo sulla politica nazionale e che spesso si limita ad un diritto di veto limitato nel tempo? Il *Bundesrat* in Austria (anche in Germania) conta - diciamolo seriamente - pochissimo. Mi domando e domando a voi tutti: è questo il destino che vogliamo riservare al Senato della Repubblica, chiamato federale ? In 1a Commissione mi sono permesso di presentare un disegno di legge che tenga conto di queste critiche e che si ispiri più al modello svizzero che a quello tedesco o austriaco, nei quali il cosiddetto *Bundesrat* ha poca rilevanza istituzionale e politica. Il nostro disegno di legge n. 24 - probabilmente perché era il primo presentato in materia - è già stato incardinato. Ringrazio il presidente della Commissione, senatore Vizzini, che nella sua relazione lo cita come l'occasione che porta la Commissione affari costituzionali ad intraprendere ancora il cammino riformatore. Uno dei punti cardine del nostro disegno di legge è quello di perseguire l'obiettivo della partecipazione regionale, senza però rinunciare all'elezione diretta del Senato federale della Repubblica e senza ridurne la rilevanza politico-istituzionale. In Germania ed in Austria i membri del *Bundesrat* sono di secondo livello, eletti in forma indiretta, rispettivamente, dai Governi regionali e in Austria dai *Landtage*, cioè dai Consigli La Svizzera, invece (insieme al Tirolo una delle più vecchie democrazie d'Europa), ha scelto la via dell'elezione diretta di ambedue le Camere da parte dei cittadini. Sia il Consiglio nazionale, cioè la Camera, che il Consiglio degli Stati, la Camera delle Regioni, sono eletti a suffragio diretto. Il mio suggerimento è di fare tesoro delle esperienze estere, sia di quelle positive che di quelle negative, di mantenere l'elezione diretta, che dà più peso al Senato. Per garantire l'espressione regionale suggerisco i seguenti principi: il primo è che i senatori facciano parte del Consiglio regionale e, rispettivamente, dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano, con diritto di intervento ed obbligo di relazione, senza però prevedere a quel livello il diritto di voto. Per rafforzare ulteriormente questo diretto collegamento con le Regioni si conferma il principio che il Senato è eletto a base regionale e, nelle Province autonome, I senatori sono consiglieri regionali eletti in aggiunta al numero già prefissato dalle leggi regionali, però nelle stesse consultazioni. Il Consiglio degli Stati svizzeri, a differenza della Germania e dell'Austria, non è né di secondo livello, né limitato nelle sue competenze, che si ispirano al bicameralismo perfetto. Vorrei far riflettere su questo aspetto. Mi sembra importante sottolineare che non si può creare, dopo decenni di aspettative finalmente evase, una Camera delle Regioni per poi conferire ad essa un ruolo completamente secondario o comunque di rilievo minore. Avevo in quest'Aula già apprezzato l'obiettivo della Lega Nord nella riforma costituzionale proposta nel 2005, poi fallita nel *referendum*. Ma con la stessa franchezza avevo criticato le attribuzioni previste per il Senato federale. Non vorrei un Senato che deve circoscrivere e limitare le competenze delle Regioni, definendo i princìpi fondamentali, senza poter incidere sulla politica nazionale. Vorrei pertanto che in Senato si inizi un percorso aperto a queste riflessioni, diverso - e lo sottolineo, in accordo con il presidente Pastore - da quello intrapreso dalla Camera. Penso che sia più giusto e più serio che il Senato stesso, non un'altra Camera, rifletta sul suo futuro e sulle competenze e sull'importanza che dovrebbe ricoprire in futuro.

Nonostante l'altissimo numero di iniziative parlamentari, le leggi approvate sono quasi tutte d'iniziativa governativa, una gran parte presentate come decreti-legge, che la Costituzione prevede come misure d'emergenza; però occupano un posto sempre più invadente e riducono il dibattito parlamentare ad una ratifica con poche correzioni. Il tutto viene ulteriormente inasprito da voti di fiducia posti con sempre più alta frequenza dai Governi. Non mi sembra affatto il caso di dover

Concludo esprimendo un convinto apprezzamento degli obiettivi di questo dibattito, di un cammino comune volto a ridurre il numero dei parlamentari e a creare la Camera per le Regioni, senza però declassarla nella sua importanza.

il momento di dire "questo lo approverò e quest'altro non lo approverò mai". Penso invece che oggi sia un momento importante per condividere un percorso comune dell'intero Parlamento. Per molti anni si è raccontato ai cittadini di quanto il federalismo fosse foriero di divisioni, odio e conflitti. All'istanza di riforma avanzata dalla Lega si opponevano scenari balcanici di sangue e morte, paventando persino l'esplosione di guerre civili quale tragico sbocco del cambiamento, se non addirittura evocando gli abissi infernali della pulizia etnica, a cui avrebbe condotto questa china. Il tempo è stato galantuomo, e la politica ha fatto giustizia delle esasperazioni di una propaganda ampiamente fuori bersaglio, sovvertendone previsioni e prevenzioni, a tal punto che oggi ci accorgiamo e ci rallegriamo di come, nei rari casi in cui i partiti superano barriere e steccati, il fattore unificante si chiami federalismo. Penso, evidentemente, alle eccezionali convergenze raggiunte in occasione del varo del federalismo fiscale e alla più ampia condivisione perseguita nell'attuale circostanza, in cui si prospetta la revisione del ruolo del Senato

preconizzò la possibilità d'intesa tra maggioranza e opposizione incentrata sulla riforma del Senato e la riduzione del numero dei parlamentari. «I toni oggi sono accesi» - dichiarò in quel frangente Roberto Calderoli - «perché ci sono le elezioni alle porte. Ma dopo il voto si può ragionare con tutti e voglio vedere chi alla fine non ci sta». In realtà, confido che si torni a discutere di federalismo e riforme condivise non solo perché sia scemata la tensione elettorale o perché il Presidente della Repubblica abbia sollecitato a lasciarsi alle spalle quel clima fisiologicamente burrascoso, ma anche e soprattutto perché in tutti è presente la consapevolezza della conquista ancora incompiuta. Ne ha convenuto recentemente anche il presidente Fini, dichiarando che «senza l'ultimo anello del federalismo istituzionale, il federalismo fiscale rischia di essere una catena alla quale manca quello più importante», e che «non c'è federalismo senza Senato federale». Ne è da sempre cosciente la Lega Nord, che nella riforma costituzionale del 2005 aveva previsto, accanto alla *devolution*, la riforma del Senato e la riduzione del numero dei parlamentari. Ne sono convinte maggioranza e opposizione che, pur tra i distinguo del caso, hanno fatto della cosiddetta bozza Violante un comune punto di partenza nell'approccio riformatore. Vorrei ricordare che già nell'aprile di quest'anno, in concomitanza con l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale,

firma del senatore Zanda, che impegnava ugualmente alla riduzione del numero dei parlamentari e a «ricercare in Parlamento l'intesa con i Gruppi di opposizione sui temi delle riforme istituzionali». Si tratta d'operare sin d'ora in quello spirito di leale collaborazione ed ampia condivisione richiamato in entrambi i documenti proposti da maggioranza ed opposizione, individuando ed affermando quanto meno il minimo comune denominatore politico che collega le due proposte. Il primo passo, in tutta evidenza, è nell'accettazione della cosiddetta il cui condiviso riconoscimento quale riferimento dell'azione riformatrice rischia, tuttavia, di risultare condizionato dalla preclusione verso altri interventi riformatori in materia di giustizia o di rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo. L'auspicio, evidentemente, è che sulle divergenze delle forze politiche prevalga ancora quella spinta al cambiamento, direi al compimento di una volontà comune e diffusa ben al di là di quest'Aula, che il federalismo già in passato ha saputo suscitare.

e debba rappresentare l'inizio di un rapporto nuovo tra le forze politiche. Questo è il motivo per cui alcuni discorsi mi sembrano un po' stonati.

È un brutto periodo. Faccio parte del Gruppo Misto, ma con la mia cultura, con il mio modo di essere di sempre; non ho certamente titolo per rappresentare una forza politica, ma voglio dare lo stesso il mio contributo.

i Padri costituenti furono capaci - questo ho cercato sempre di insegnarlo ai giovani della mia scuola - di sedersi al tavolo e scrivere insieme delle regole. Uomini di cultura cattolica, di cultura marxista e di cultura liberale trovarono un meraviglioso equilibrio nel nostro documento costituzionale. Noi dovremmo ricordarlo questa sera invece qualcuno voglia strumentalizzare questo dibattito per raggiungere scopi di ordine privatistico come forza politica.

impone decisioni rapide, pur nella salvaguardia assoluta del dibattito parlamentare e della democrazia. Bisogna però avere, caro ministro Calderoli, un progetto globale che coniughi questa riforma con il federalismo, con la riforma delle autonomie locali: questo è un aspetto da concordare tra le forze politiche in un documento.

quello che abbiamo favorito negli ultimi anni, cioè l'egoismo tra i livelli istituzionali. Non possiamo creare la Repubblica dei patti attorno ai tavoli nei quali si concorda tutto. Dobbiamo creare una Repubblica delle regole nella quale ogni livello di potere deve rispettare le regole. Ecco perché io credo che tutto debba anche partire, caro Ministro, dalla legge elettorale: la madre di tutte le battaglie. La legge elettorale è il cancro di questo sistema. Anche se ho poca esperienza di questo Parlamento, mi sono reso subito conto che la legge elettorale uccide la libertà del parlamentare, la elimina totalmente. Bisogna assolutamente ridare al popolo la libertà di scegliere e ridare dignità al parlamentare. Ecco perché è necessario che

Signor Presidente, illustri senatori, le riforme istituzionali oggetto di possibili leggi sia di rango costituzionale sia ordinario sono una materia nobile che personalmente vorrei avesse sempre una propria valenza assoluta, non fosse cioè condizionata dalle contingenze politiche del momento. Ma poiché così non è (e a maggior ragione non può esserlo oggi che viene portato un evidente attacco frontale a chi ha ricevuto dal popolo il mandato di governare), lascio volentieri ai nostri Capigruppo la prerogativa di trattare degli scenari politici sul cui sfondo parliamo di riforme. Scelgo - ho scelto da più anni - di occuparmi solo del contenuto delle possibili o auspicabili riforme. Lo faccio nient'affatto a titolo individuale,

documento e divergendo in parti essenziali da progetti, bozze o proposte, delle quali troviamo allo stato condivisibile, più che altro, una parte dell'indice, confermiamo di considerare positiva e degna di essere promossa una evoluzione del sistema istituzionale orientata verso questi chiari ed espliciti obiettivi: ragionevole diminuzione del numero dei deputati e dei senatori, perché si contemperi lo snellimento delle compagini parlamentari con la indispensabile rappresentanza delle molteplici realtà sociali e territoriali; valorizzazione della risorsa costituita dal bicameralismo, con superamento del bicameralismo perfetto, mediante Camera alta e Camera bassa differenziate per composizione, forse anche per rapporto di fiducia politica con l'Esecutivo, ma entrambe elette a voto diretto dal popolo ed esercenti piena sovranità legislativa democratica; terzo, rilanciata e virtuosa interazione tra rafforzati poteri del Governo scelto dagli elettori e potenziate facoltà delle Camere e del singolo parlamentare; quarto, revisione del sistema giudiziario e dei suoi organi di regolazione, nel quadro di un recuperato equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, nello Stato di diritto e nel rispetto e nel rispetto della sovranità dei cittadini democraticamente espressa; quinto, incisiva revisione del sistema delle autonomie con decisa e reale semplificazione dei livelli di governo regionale e locale, perché siano promosse la partecipazione dei cittadini e la valorizzazione delle identità nella logica dell'unità nazionale e della più responsabile coesione sociale. Sulla base di questi punti, che io ed altri ci onoriamo di aver sostenuto con coerenza intellettuale fin dal tempo delle nostre legislature da deputati, ci apriamo al più schietto e libero confronto, senza alcuna rigidità di schieramento ma altrettanto alieni da dialoghismi di maniera, entrambe di troppo vecchio costume appartenenti ai riti della manovra politica, non certo al profondo e durevole culto delle istituzioni. Ci auguriamo, poiché - fino a prova contraria - stiamo parlando nell'odierna Camera Alta della Repubblica, che il Senato emetta in questa occasione e su questa materia non una eco o un brontolio riflesso, ma un proprio, vigoroso, moderno contributo originale e un segno forte ed autorevole della propria creativa esistenza.

nei lunghi anni in cui si è svolto, ha portato il comune sentire dei cittadini da un livello di indifferenza ad uno di attenzione propositiva, oggi purtroppo di quasi incredula rassegnazione. Rimane comunque forte e viva la consapevolezza della necessità di un complesso insieme di riforme, al quale potremmo sottrarci - in maniera consapevolmente irresponsabile lasciando andare alla deriva l'intero Paese e il suo futuro. Non saranno gli altri, non sarà l'Unione europea, a fornirci i moderni strumenti istituzionali dei quali abbiamo assoluto bisogno, siano essi riguardanti la legislazione ordinaria o costituzionale.

come magari preferisco, più modestamente, alle assemblee dei lavoratori, ai convegni degli imprenditori, alle classi sociali che oggi maggiormente soffrono del peso derivante dai lacci con i quali si è

ripeto - la nostra attenzione si deve rivolgere soprattutto a questo secondo ambito. Vi ricordo, colleghi, volendo portare alla vostra attenzione soltanto uno tra i molti esempi possibili, quello delle relazioni sindacali e sociali, che in alcune delle Regioni nelle quali la crisi economica ha prodotto ripercussioni molto profonde, esse si sono intrecciate in maniera assolutamente innovativa. Qui si assiste ad imprenditori e maestranze che, attraverso i loro rappresentanti, le loro associazioni, i loro sindacati (possiamo non ricordare gli anni di assoluta conflittualità?) stanno superando ogni tatticismo di maniera a strenua difesa del posto del lavoro, nella piena consapevolezza dell'importanza della coesione quale unico strumento attraverso il quale permettere la sopravvivenza delle aziende e delle famiglie. Non ci chiedono miracoli - sanno che le risorse e i mezzi a disposizione del Governo sono limitati - ma ci chiedono coerenza nell'assunzione della nostra parte di responsabilità; di adempiere, come loro stessi hanno fatto, il nostro compito per una riforma complessa e profonda del Paese. Vogliono sapere dove e in quale modo vengono spesi i loro soldi, vedere l'attuazione del federalismo fiscale, la soppressione della pletora di enti pubblici soffocanti e costosi, la riduzione dei gangli della politica, il potenziamento dell'azione legislativa e la riorganizzazione e la trasformazione dell'azione giudiziaria. I cittadini oggi, questi cittadini, guardano al Parlamento e alla magistratura come a dei mostri tentacolari che si autoalimentano o, peggio, che si alimentano grazie alle loro stesse sofferenze, all'interno di una competizione che li lascia esterrefatti. Mi chiedo quale enorme effetto potrebbe avere, ai fini delle libertà civili ed economiche, una riforma profonda della nostra Costituzione realizzata con ampio consenso parlamentare; quali potrebbero essere gli effetti sull'incremento della fiducia dei cittadini, sulla propensione agli investimenti, sulla motivazione dei giovani ad assumere responsabilmente e con entusiasmo le redini del futuro. Dovremmo dedicarci a queste considerazioni, a quanto al di fuori di queste Aule ci viene chiesto, a quanto viene auspicato, e che funzione sociale, economica, civile in generale potrebbero avere potrebbero avere delle nostre scelte fatte con decisione, rapidità e coesione. Oggi non basta più fare il gioco delle parti. Nel dibattito odierno hanno assunto una valenza condivisa molte delle modifiche costituzionali approvate nel 2006 e cassate da un *referendum* popolare per il quale la contraddizione ha purtroppo avuto la meglio sulla progettualità. E' un obiettivo possibile, probabilmente l'unico perseguibile, se non vogliamo renderci responsabili di un immobilismo istituzionale che non lascerebbe scampo al Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'invito rivolto a tutti dal Presidente della Repubblica per avviare un dialogo costruttivo è stato saggiamente accolto dal Senato, e credo che il dibattito di oggi su mozioni dai contenuti molto simili possa dare agli italiani, in un momento certamente non sereno per la politica, la speranza che attraverso un risorto spirito costituente, per quanto timido, le forze politiche presenti in Parlamento vogliano veramente riprendere quel percorso di riforme più volte fallito per vari motivi. Saremmo ingenerosi se non avessimo l'onestà intellettuale di riconoscere che se la Lega non avesse incalzato sul processo delle riforme in senso federale, noi oggi probabilmente non ci porremmo ancora il problema di una riforma più compiuta, a partire dai temi su cui nel tempo si è già trovata una forma di convergenza: sulla differenziazione dei compiti delle Camere con l'introduzione del Senato federale, sulla conseguente riduzione del numero dei parlamentari, sul riequilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento. Affrontare oggi il tema delle riforme non è allora una sorta di prova tecnica di dialogo (che pure è di grande importanza), ma è un dovere preciso quanto improrogabile di questo Parlamento che, anche a seguito dell'approvazione della norma sul federalismo fiscale, ha il dovere di disegnare regole certe a garanzia dell'unità della Nazione in una Repubblica a base federale. Certamente, quella che era la cosiddetta bozza Violante, oggi riproposta alla Camera da Sesa Amici e da Italo Bocchino, può rappresentare un punto di partenza utile per riaprire un dialogo che pretestuosamente o con superficialità si arenò nella scorsa legislatura. Partiamo quindi, come spesso ripetiamo, da ciò che unisce, dall'esigenza di dire basta al cosiddetto bicameralismo perfetto, dando al Senato federale quella funzione che oggi deve avere, perché ormai il federalismo non è più un obiettivo politico da conseguire, ma è legge ed è dunque giusto e corretto che le espressioni dei territori, fino ad ora rappresentate solo nella Conferenza Stato-Regioni, con tutti i limiti che la stessa ha rispetto agli aspetti decisionali, trovino nel Senato federale la sede giusta per assumersi, davanti allo Stato e all'interno del Parlamento, le proprie responsabilità. Trovo che questo sia un aspetto di fondamentale innovazione nei riguardi dei territori in generale, e dei cittadini più in particolare, che debbono essere messi sempre più in grado di saper individuare e riconoscere le responsabilità per regolare poi i loro comportamenti elettorali. Il problema non sarà solo quello della riduzione del numero dei senatori, quanto le modalità di elezione. Se si vuole assicurare una certa funzionalità al sistema delle autonomie non può ignorarsi la previsione che i senatori siano eletti in parte dai consigli regionali e in parte delle autonomie locali, perché si rischia di non assicurare la richiesta omogeneità funzionale e amministrativa. Si potrebbe immaginare un Senato federale composto direttamente con rappresentanti delle Giunte regionali, nel qual caso, in assenza di senatori eletti, non avrebbe più senso diminuire il numero di parlamentari della Camera dei deputati, ma evidentemente è solo un'ipotesi di lavoro. Oggi quel che importa è affermare il principio dell'assoluta necessità di diversificare le funzioni delle due Camere, che eserciterebbero ambedue la funzione legislativa solo in occasione di leggi costituzionali, elettorali, in materia di organi di governo ed enti locali, di funzioni dello Stato, di informazione ed emittenza radiotelevisiva, ratifica di trattati, amnistia e indulto. Tra le mozioni in discussione questi punti sono indubbiamente condivisi e possono rappresentare un buon punto di partenza per riprendere, in maniera *bipartisan,* il tema delle riforme di grande momento. Non vorrei tuttavia rimanere nell'ambito di una ovvia adesione a una riforma minimale. Parlare di riforme significa anche affrontare finalmente due temi che con coraggio sono presenti nella mozione del Popolo della Libertà: l'avvio della discussione sul rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo, nell'ambito di una coerente e riequilibrata revisione della forma di Governo, e una riforma delle norme di rango costituzionale che sovrintendono al funzionamento del nostro sistema giudiziario. Sono due temi forti, ma fondamentali per dar vita non ad una Terza Repubblica, ma ad una nuova Repubblica, quella che era già *in nuce* addirittura nei dibattiti in fase costituente (ricordiamo Calamandrei e Costamagna) e che fa parte della storia italiana del

indicava - già negli anni Sessanta - l'esigenza di superare i contrasti drammatici del passato per cercare un'intesa riformatrice capace di superare le differenze tra posizioni di centro, di destra e di sinistra. E poi l'esperienza di un gruppo di dirigenti democristiani, e ricordiamo ancora Crisafulli, La Pergola, Augusto Del Noce, e quella dello stesso Craxi, che ebbe il merito di sdoganare il dibattito sulla necessità di una grande riforma. Ma per me, di cultura tradizionale di destra mai rinnegata, non può essere messa nell'oblio la proposta politica del 1979 di Almirante e Romualdi presente in una loro mozione parlamentare, né tantomeno l'intenso dibattito e la costruzione del progetto costituzionale di Repubblica presidenziale. Tutto questo non posso e non voglio dimenticare: appartiene alla mia storia politica, che indubbiamente è poca cosa rispetto al grande tema delle riforme, riforme, che va affrontato con urgenza perché siamo ormai di fronte a quello che Panebianco ha acutamente immaginato essere il tramonto del bipolarismo. Un Parlamento che intenda essere responsabile nei riguardi del popolo sovrano non può accrescere l'ingovernabilità e l'instabilità ma ha il dovere, dopo tanti - troppi - anni di dibattiti inconcludenti, di affrontare e risolvere il grande tema della forma di Governo. La già ricordata bozza Violante, con il suo rafforzamento, sia pur lieve, dei poteri del *Premier* che può nominare e revocare i Ministri è sufficiente per dare una risposta? Personalmente ritengo di no. L'elezione diretta del Capo dell'Esecutivo con il contrappeso del rafforzamento dei poteri del Parlamento sarebbe la conclusione giusta e coerente di un percorso iniziato felicemente con l'elezione diretta dei sindaci e quindi con l'affermazione forte della partecipazione popolare. Quanto al secondo tema forte, la giustizia, sono anch'io convinta che ormai una riforma radicale non sia più procrastinabile. È un problema di democrazia reale, di tutela dei diritti, di assunzione di responsabilità dalle quali non esiste in democrazia che qualcuno o una categoria possa essere esonerato. Non sono un giurista, ma da cittadina conosco una norma generale: la giustizia deve anche apparire, oltre che essere, giusta. Francamente, sapere che può esistere una magistratura democratica, una magistratura indipendente, una magistratura che si rifà alla Costituzione non dà certamente tranquillità al cittadino; credo debba esserci una magistratura lontana dalla politica, che sappia recuperare fino in fondo la dignità del suo ruolo e della sua missione a difesa a difesa dei diritti del cittadino. In quella magistratura, noi vogliamo continuare a credere. Una magistratura forte della dignità del suo delicatissimo compito, lontana dai riflettori ma rigida e discreta ad un tempo, rispettosa anche del più elementare dei diritti del cittadino comune, comune, quello a non essere sbattuto in pasto a stampa e *media*, avendo egli diritto alla presunzione di innocenza e non, invece, a quella di colpevolezza. Per questi motivi, per la mia tradizione di cultura politica, per i sentimenti che nutro nei riguardi di questo processo riformatore che è troppo lungo ma che può veramente avviarsi ad una conclusione, mi auguro, Presidente, che vi sia un documento comune che riesca a riassumere, in sintesi, quelle linee di indirizzo che sono state efficacemente ritrovate in tutti i documenti qui presentati, ma soprattutto mi auguro che questo Parlamento voglia finalmente dare le risposte che tutto il popolo merita e aspetta da troppo tempo.

ma sembra mancare una riflessione sulla legge elettorale rispetto al *vulnus* introdotto dal 2006 nel rapporto tra cittadini ed elettori e questa assenza inficia anche i ragionamenti che possiamo fare su tutte le altre architetture istituzionali. Un conto è un rapporto che sgorga da una conoscenza diretta e reciproca e da una possibilità di valutazione tra singolo cittadino e candidato; altro conto è il rapporto anonimo che abbiamo costruito con queste anomale e lunghissime liste bloccate, la cui lunghezza non trova riscontro in nessuna altra democrazia contemporanea, con uno svilimento del principio di sovranità popolare affermato solennemente dall'articolo 1

e non aveva mai conosciuto né questa aberrazione delle liste lunghissime e neanche gli effetti negativi molto forti (che abbiamo visto poi esplodere con Tangentopoli) legati all'uso del sistema delle preferenze e al costo delle campagne elettorali. La legge elettorale del Senato, prima della forzatura del 2006 che l'ha praticamente clonata - regione per regione - sul modello nazionale, ha avuto sempre nella storia del Parlamento democratico

dall'esito referendario, essendo più figlia diretta del quesito referendario che verteva sul Senato, produsse una legge di gran lunga migliore al Senato rispetto alla Camera dei deputati. Infatti, alla Camera, il meccanismo della doppia scheda finiva per separare, nella competizione proporzionale, coloro che erano uniti nella competizione maggioritaria, tanto è che per diversi anni

posizione anche in un ordine del giorno, a sua prima firma, votato dal Senato il 16 gennaio 2001. In esso egli richiamava la necessità di ripristinare il collegio uninominale. Ricordo la formulazione di quell'ordine del giorno, presentato da Leopoldo Elia e approvato in quest'Aula, che così recitava: «(...) ritiene che si debbano preferire una forma di Governo ed una legge elettorale che facciano emergere da una sola consultazione degli elettori la maggioranza parlamentare e l'indicazione del Presidente del Consiglio, in modo da incorporare la scelta del leader nella scelta della maggioranza»

sul ripristino puro e semplice della legge previgente. Certo, poi potremo fare anche di meglio, perché esistono tante altre soluzioni, ma oggi dobbiamo solo fare un elenco dei temi e in questo elenco non può non essere ricompreso quello del ripristino del collegio uninominale,

la crisi economica in particolare impone un'accelerazione sulle riforme. I cittadini ci chiedono sempre più dibattiti tranquilli e sereni come questo. I cittadini ci chiedono risposte e, una volta tanto, di smetterla con risse che non conducono da nessuna parte.

Noi riusciamo nella straordinaria impresa di spendere ogni anno 800 miliardi di euro, laddove quest'anno ne entrano solo 720 miliardi. Quindi, vi è un buco di 80 miliardi. Questa è la situazione dopo la crisi

È evidente che si tratta di una situazione paradossale e impossibile. Oppure, se preferite, dovremmo fare tre «finanziarie Prodi» da 25 miliardi di euro, più una normale da

Dunque, di fronte a una realtà che i numeri esprimono in maniera così chiara, è evidente a tutti che

Dovremmo metterci tutti una mano sulla coscienza per porre mano pesantemente alla questione, perché è evidente che altrimenti si crea un danno alle nostre imprese, alle nostre famiglie e, come minimo, facciamo scappare gli investitori esteri.

uno studio dell'Agenzia delle entrate del 2006 ha elaborato un'analisi regionalizzata dell'evasione fiscale. In Lombardia, che è la regione più virtuosa, sfugge al fisco il 13 per cento dell'imponibile. In

per ogni 100 euro dichiarati, ne spendono 106, cioè 6 euro in più. Guarda caso i conti tornano alla lira o, se preferite, all'euro:

48 euro in più. Guarda caso i conti tornano all'euro: per ogni 94 per cento di imponibile che sfugge, il 50

L'unico modo per risolvere una situazione così compromessa è fare riforme vere, pesanti, incisive e attuare il federalismo fiscale. Solo così riusciamo a mettere i conti a posto, ed è anche opportuno farlo in fretta perché, vista la situazione dei conti pubblici, rischiamo che tra un po' sia troppo tardi. *(Applausi

che il Senato chieda al Governo di essere sollecitato a fare quello che il Senato già dovrebbe fare da solo. È come se

questo attorcigliarsi in una spirale non comprensibile. Peraltro, anche nella mozione che chiede al Senato di impegnare se stesso a fare una cosa, trovo un elemento di perplessità: il Senato fa

è molto affezionato alla Carta costituzionale e non ritiene quindi che i problemi

Alcune cose sicuramente possono e devono essere fatte: il collega Pardi ne ha citate diverse,

che ha introdotto profonde storture nella nostra produzione legislativa, nonché il divieto di rientro nei ruoli, alla fine del mandato parlamentare, dei magistrati eletti. Una cosa però non vogliamo che venga toccata, vale il Titolo IV della Costituzione, che attiene all'ordinamento giurisdizionale e alle norme sulla giurisdizione.

giustizia, dimostrando però una pervicace ostinazione a litigare con la Carta costituzionale.

con il lodo Alfano, dichiarati anch'essi incostituzionali; ora ci volete provare con il processo breve, manifestamente e clamorosamente incostituzionale! Noi abbiamo un'avversione totale a questi vostri tentativi di avvicinamento alla giustizia; quando ne parlate ci viene l'orticaria. Temiamo quello che potete riuscire a fare nel distruggere un sistema che noi invece vogliamo difendere.

con i vostri interventi demolitori per proteggere «un monarca assoluto», come ha detto un alto rappresentante della vostra maggioranza. Siamo stufi dei monarchi assoluti: vogliamo cittadini uguali dinanzi alla legge, e difenderemo la nostra Costituzione contro la vostra arroganza e la vostra violenza nel legiferare.

che è stata assunta e la volontà che essa esprime di un dibattito e delle possibili conclusioni sulle necessarie riforme costituzionali. Mi auguro che a questo si arrivi sollecitamente, perché lo ritengo necessario onde porre termine alla consuetudine di attribuire le degenerazioni e le insufficienze della politica alle mancate riforme costituzionali. Mi auguro che il nostro lavoro, e soprattutto il lavoro di quelli che saranno addetti a preparare i testi costituzionali, sia ispirato ad una sobrietà costituzionale.

ha guidato il nostro Paese in trasformazioni fondamentali, tanto economiche quanto politiche. Ritengo che se non avessimo avuto mancanza di sobrietà costituzionale nei precedenti tentativi di modificare o di fare le riforme necessarie alla Costituzione, non avremmo avuto la bocciatura del progetto nel *referendum* tenuto tempo addietro. Vorrei auspicare che né formalmente né surrettiziamente la Costituzione incrini il principio dell'unità nazionale su cui essa si fonda. Mi auguro altresì che il cosiddetto rafforzamento delle posizioni del Primo ministro non significhi introdurre una forma di presidenzialismo nella nostra Costituzione, cioè non significhi trasformare una Repubblica, che è e deve restare parlamentare, in una Repubblica presidenziale. Non dobbiamo, dunque, cedere a tentativi del genere, come del resto mi è parso di sentire anche in alcune dichiarazioni rese in quest'Aula. Mi auguro altresì che le modifiche non tocchino gli equilibri tra i poteri quali sono stati definiti nella Carta costituzionale vigente; caso mai, attraverso forme adeguate, se ne realizzi il più adeguato e corretto funzionamento. Mi auguro altresì che a tutti coloro che lavoreranno direttamente a queste modifiche sia chiaro che non basta affermare che non si deve modificare la prima parte della Costituzione; ma si deve avere sempre chiaro dinanzi a sé che anche modificando la seconda parte della Costituzione si può, in qualche modo, incidere sulla prima parte, dichiarata non riformabile ed accettata da tutti. Faccio questa dichiarazione - mi consentiranno i colleghi - con l'emozione e la convinzione con cui votai il testo costituzionale nel 1948.

lo faccio in nome non di un blocco sociale che include la mafia, ma in nome di un'altissima tradizione culturale, che è stata al centro ed è stata il perno nella preparazione, nella discussione e nella formazione della Carta costituzionale che ha guidato l'Italia in questi sessant'anni.

alla scuola di Manin. Un'altissima tradizione culturale che poi significa De Gasperi e - perché no, caro senatore Macaluso? - anche Fanfani e Moro, da lei citati nella sua dichiarazione

benché oggi sia un po' dispersa e un po' indebolita, deve essere presente in questa azione che noi intraprendiamo di modifiche relative e necessarie di riforma costituzionale. finestra") *(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ora che le riforme sono iscritte all'ordine del giorno del dibattito politico (perché giovano al Paese, non a qualcuno), cui lavora una riforma, specie quando influisce sugli assetti fondamentali dello Stato, può rivelarsi più importante del suo stesso contenuto. Infatti, tanto per citare l'esempio più eclatante degli ultimi tempi, mi chiedo, con riferimento alla riforma del Titolo V voluta dall'Ulivo e al federalismo fiscale introdotto dal centrodestra: è sicuro che il federalismo fiscale, senza una forma di Governo basata sul voto diretto degli elettori, alla fine non susciti una competizione politica per territori, anziché per grandi idee, valori e forze politiche nazionali? In questo senso, il riferimento alle polemiche che sempre suscitano le dichiarazioni del ministro Bossi è alquanto significativo. La risposta l'ho cercata e l'ho trovata ripensando a quel complesso del tiranno, richiamato anche nell'intervento del senatore Colombo, che spinse il costituente del 1948 a controbilanciare i poteri del Presidente del Consiglio con quelli del Capo dello Stato e di un Parlamento bicamerale. Nello Stato post-monarchico e romanocentrico del tempo, infatti, un sistema di tipo democratico non poteva che trovare il suo punto di rottura là dove con il fascismo, in effetti, lo trovò anni prima: al centro, nel luogo dove la concentrazione di potere era massima e da dove qualcuno (un nuovo Primo ministro in vena d'avventure) poteva partire per rompere il circuito democratico e far deragliare la giovane e fragile democrazia verso approdi autoritari. Quello del 1948, insomma, è un sistema di Governo e di equilibrio di poteri costruito contro qualcuno: il Primo ministro. Ma oggi la sovranità non si esaurisce nello Stato; essa si colloca in più punti dell'ordinamento. Oggi il potere vero si trova disperso in più sedi, in più mani, in più istituzioni.

agli organismi internazionali ed europei, con la perdita di sovranità dello Stato unitario verso l'esterno (penso alla Comunità europea, per non parlare delle sedi internazionali), agli stessi tribunali internazionali, alle stesse autorità di garanzia, ai partiti politici, ai sindacati, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni non governative, alle associazioni delle comunità di immigrati, ai movimenti di genere, ai gruppi di pressione, alle associazioni di volontariato, alla stampa, alla tv, alla Rete, alla comunicazione satellitare (tutti i mezzi di comunicazione esercitano comunque quote di sovranità). Oggi che il federalismo costituzionale, istituzionale e fiscale ha creato, di fatto, un sottosistema di governo parallelo e ramificato come quello nazionale; oggi che tutti i politologi e gli studiosi parlano di una democrazia che ha assunto forme policentriche e persino poliarchiche, collega Pardi, trovo davvero poco coerente alla realtà e considero una tesi arretrata dal punto di vista culturale, lontana dalle esperienze delle democrazie governanti, quella che sostiene una possibile deriva plebiscitaria affermando che qualcuno, all'improvviso, possa impossessarsi di tutto. Oggi è veramente assurdo affermare che il punto di rottura del nostro sistema democratico possa essere l'autoritarismo di qualcuno e non, piuttosto, la disgregazione di qualcosa. Oggi il rischio vero che corre la nostra democrazia non è che qualcuno, sentendosi un monarca assoluto, si impossessi di tutto; il rischio vero è che la cosiddetta democrazia diffusa, di per sé positiva, alla fine, se non accompagnata da limiti unitari invalicabili e dalla scelta diretta di chi governa, possa sgranarsi a tal punto da perdere ogni contatto con il suo centro, determinando la disgregazione del corpo della Nazione. Il rischio vero, che denuncio, è che, dopo una prima fase nella quale al confronto tra i grandi partiti nazionali si sostituisca quello tra i partiti dei territori, segua una seconda fase nella quale si fa più forte l'eventualità che i pezzi se ne vadano per conto proprio. Una Carta costituzionale si difende, caro senatore Colombo, applicandola, ma modificandola secondo le norme che essa stessa prevede. Ebbene, vedo un rischio nella democrazia contemporanea sempre più sgranata, mediatica, liquida e virtuale. Colleghi, non credo siano sufficienti l'azione centripeta di una semplificazione bipartitica della legge elettorale e un Governo con qualche potere in più, ma sempre figlio del modello parlamentare. Per evitare che l'azione centrifuga si snodi in mille centri di potere, oggi occorre proteggere la tenuta unitaria della nostra Repubblica. Non credo che alla competizione per ideali si possa sostituire quella dei territori; non credo quindi che i correttivi di cui alla bozza Violante, motivati da una diffusa diffidenza verso il voto diretto degli elettori,

C'è stato, durante la seconda Repubblica, un grande momento di tensione unitaria durante il quale si cercò di rinnovare il patto costituente attraverso una Costituzione pensata. Risalgo allo spirito costituente del 1948, perché il modello è quello; solo che una Costituzione moderna, di oggi, per la democrazia contemporanea, non può essere più pensata contro qualcuno, bensì contro qualcosa: il pericolo della disgregazione. Mi riferisco alla Commissione bicamerale D'Alema-Berlusconi: più che riforme al ribasso, in quella Commissione bicamerale unitaria si cercò di dare una risposta parlando di un Governo forte, di un Parlamento forte, di un sistema di garanzia forte e di un federalismo forte. Ritengo che all'interno di tale equilibrio si possa trovare quella via maestra in grado di fare del nostro Paese una vera democrazia governante. Grazie *(PdL)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, mi accingo a questo intervento con la speranza

per lasciarne traccia nei verbali dei lavori del nostro Parlamento, senza che si abbia mai la capacità di vivere una stagione importante di cambiamento. Dopo la riforma del Titolo V, del 2001, è iniziato il processo delle riforme possibili con legge ordinaria. Tra tutte voglio ricordare il federalismo fiscale,

alle autonomie locali, difficilmente avremo una forma di federalismo vero basato solo sulle compartecipazioni. Se non faremo questo, lo dico perché credo che tutti dovremmo avviare una riflessione, avremo la metà dei governi del Paese che vivrà senza un principio della democrazia: «*no taxation without representation»*, perché vivendo di compartecipazioni si vive di responsabilità parziali. Rischiamo, però, di creare un mostro giuridico nel modo di essere del nostro Paese se adesso non mettiamo mano al cambiamento della Costituzione. Non ci può essere assetto federale dello Stato

paura: Giuliano Amato diceva che i Costituenti non l'avevano affrontato perché avevano il complesso del tiranno; ho l'impressione che questo complesso viva e attraversi ancora il sistema politico. Vorrei però che si riflettesse e che prendessimo tutti atto del fatto che dopo il trasferimento di poteri e competenze dello Stato verso livelli di territoriali di Governo più vicini ai cittadini - le Regioni, i Comuni, le Province - anche con l'elezione diretta dei vertici di questi enti, il sistema risulta assolutamente sbilanciato: l'Esecutivo nazionale è debole e la democrazia parlamentare è soltanto un esercizio verbale del quale spesso ci riempiamo la bocca quando affrontiamo i temi L'Italia è un Paese dove la democrazia parlamentare è forte, forse è la democrazia parlamentare più forte e radicata di tutta l'Europa occidentale - quella che ha una storia di democrazia il processo legislativo sta funzionando con uno squilibrio dei poteri che si è creato, un po' come succede quando un'arteria non porta più il sangue direttamente al cuore e si formano dei circuiti paralleli che lo fanno. Quel cuore, però, non funziona bene, come non funziona bene il nostro sistema, poiché oggi vige un modo di legiferare che, a prescindere da chi governa, mortifica la democrazia parlamentare. Per cercare di rispondere alla domanda pressante di rapidità di legislazione e di decisione di una moderna democrazia governante,

decreti-legge, voti di fiducia, maxiemendamenti, ordinanze di protezione civile, uso abnorme delle deleghe ed altri simili artifizi sono le risposte che oggi si danno alle esigenze della società e dell'economia, i Governi cercano di rispondere in tempi brevi violando le regole della democrazia parlamentare. Stiamo creando dunque un sistema, in cui ci stiamo assestando, che vìola le regole della democrazia parlamentare per dare delle risposte in tempo reale. A questo bisogna saper mettere mano se vogliamo davvero cambiare, mutando il ruolo dei due rami del Parlamento senza mortificarne alcuno. Io mi rifiuto di chiamare «Senato delle Regioni» una cosa che non conosco. Io dico che ci vuole un ramo del Parlamento che mantenga il contatto con il territorio

costituzionale tutta una serie di conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni perché non c'è un ramo del Parlamento che può essere la stanza di mediazione politico-istituzionale di questi temi. Com'è pensabile che si possa sviluppare un federalismo se non ci apriamo a questo tipo di di cambiamenti? Questo è lo sforzo che dobbiamo saper fare: ritrovare la strada di un Paese che abbia un Governo forte, come sono forti i Governi locali. Non m'interessa in questo momento l'elezione diretta: c'è la legittimazione diretta del Presidente del Consiglio perché il nome dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio è oggi scritto nel simbolo dei partiti e, quindi, nella scheda elettorale. È una legittimazione diretta, ma ci vuole un Governo. Il tema non è soltanto nominare e revocare i Ministri, ma anche come dare alla società che cambia le risposte in tempo reale perché, se viene la ripresa economica, i Paesi che prenderanno il vento della ripresa sono quelli che hanno il migliore apparato statuale, la migliore organizzazione sul territorio e il migliore funzionamento delle istituzioni. Questo dobbiamo Concludo dicendo che questo sforzo va fatto cercando le forme più ampie di collaborazione in Parlamento. Mettiamo da parte gli errori del passato e con essi sia l'uso della maggioranza semplice per vincere sulla minoranza sia il diritto di veto della minoranza che, per portare al*referendum*, ha cercato di fermare lo sforzo della maggioranza. Ci vuole una mediazione alta, seria, forte; per una volta pensando non tanto ai nostri partiti, ma alla vita della nostra Repubblica, che è di tutti i partiti e senza la quale non ci sarebbero i partiti. Questa è la lezione che abbiamo ricevuto dai Costituenti in un difficilissimo momento in cui bisognava rifondare la democrazia in questo Paese. Tutti i pesi e contrappesi vennero in una Repubblica che nasceva che nasceva dalle ceneri di una monarchia, in una democrazia che nasceva da una dittatura. Oggi dobbiamo ritrovare gli equilibri persi tra i poteri dello Stato. Si tratta di un compito non meno difficile

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo sia ormai sotto gli occhi di tutti che il nostro Paese ha bisogno delle riforme. Proprio per questo considero particolarmente importante discutere in Senato le diverse mozioni che i Gruppi hanno presentato, e che al proprio interno contengono impegni simili. Il dato significativo è che si parte, infatti, da una base comune. Una per tutte: la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto, che non significa affatto indebolire, ma rafforzare il ruolo del nostro Senato. Sono impegni che noi, come Gruppo della Lega Nord, portiamo avanti da sempre e siamo felici che si possa giungere ad una sintesi tra diverse posizioni politiche, nell'interesse esclusivo di tutti i cittadini. Era da tanto, forse da troppo tempo che, a parte le dichiarazioni di intenti un po' rituali, non si faceva qualcosa di concreto. Dobbiamo riconoscere, invece, alle forze politiche responsabili qui rappresentate di avere intrapreso la strada giusta. La nostra gente vuole le riforme; noi le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale e le vogliamo realizzare senza divisioni e con il contributo di tutti. Vogliamo far sì che non si continuino a cambiare le regole del gioco appena si apre una nuova legislatura. È per questo che siamo disponibili al dialogo con coloro che lo vorranno. Dobbiamo dare tutti quanti noi un segnale: superare le barricate ideologiche che non portano da nessuna parte. Le riforme vanno assolutamente affrontate senza pregiudizi e senza esasperare gli scontri o i toni del dibattito. Lo abbiamo scritto anche nel testo della mozione di cui sono fronte, impegna il Governo: ad incoraggiare, con spirito di leale collaborazione, un confronto parlamentare sui temi delle riforme istituzionali, per giungere alla necessaria approvazione di un testo condiviso dalla più ampia maggioranza Purtroppo, il processo di riforma costituzionale è già stato diverse volte esposto al pericolo di un'interruzione o di una dispersione lungo percorsi inconcludenti e paralizzanti. Ecco perché il tempo delle chiacchiere è finito. Questa volta si fa sul serio. Il Governo ha avuto un mandato chiaro dai cittadini. Dobbiamo lavorare di comune accordo per implementare quel processo riformatore di cui si sente tanto la necessità: prima tra tutte la riforma del Parlamento, con la riduzione del numero dei suoi membri ed il superamento del bicameralismo perfetto. Constatiamo, infatti, ogni giorno le lungaggini del procedimento legislativo, dovute all'attuale meccanismo di doppia lettura, prima di giungere all'approvazione di un medesimo testo di una proposta di legge. L'esperienza ci suggerisce, quindi, soluzioni che superino gli inconvenienti del sistema vigente. I procedimenti legislativi dovranno dunque essere improntati all'efficienza, alla snellezza e alla rapidità nella decisione. Occorre, inoltre, interrogarsi sull'opportunità, di fronte ad una società sempre più complessa e ad una maggiore articolazione dei livelli di governo, di procedere ad una riforma del nostro Parlamento che assicuri una integrazione della rappresentanza, prevedendo ad esempio la trasformazione della Camera alta in Senato federale. Un altro tema di rilievo, che abbiamo voluto porre all'attenzione dell'Assemblea, è la revisione della forma di Governo, nel senso che vorremmo promuovere l'avvio di una discussione su un rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo, preservando comunque l'equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. A mio avviso, il rafforzamento del ruolo dell'Esecutivo non è e non deve essere declinato come un rafforzamento a danno delle Camere. L'obiettivo, al contrario, è quello di aver un rapporto più stretto e autorevole con il Governo, per un sistema parlamentare più efficiente e moderno, in grado, più che di paralizzare l'azione dell'Esecutivo, di controllare e verificare puntualmente la sua concreta attività. Infine, con la mozione PdL-Lega, vorremmo impegnare il Governo a porre in essere un'azione di riforma delle norme che sovraintendono il funzionamento del sistema giudiziario. Anche su questo tema, mi auguro che si possa svolgere un dibattito costruttivo tra tutte le forze politiche, che possa condurre ad ipotesi condivise, quanto mai necessarie. Vorrei, infatti, che la consonanza di intenti e di indirizzi tra i due schieramenti sul tema delle riforme istituzionali portasse ad aprire una vera stagione riformatrice. Voglio essere ottimista sulla possibilità che si giunga ad un confronto fruttuoso e veramente *bipartisan* per rendere più adeguate le istituzioni alle attese dei cittadini. Gli stimoli, come vedete, sono molti e le prospettive di sviluppo molteplici. Su questa via dobbiamo impegnarci tutti, con unità di intenti, per il bene di un Paese ancora troppo assistenzialista e centralista. È ora di far seguire alle parole anche i fatti. Non bisogna perdere l'occasione per cambiare e migliorare il nostro Paese.

penso che nell'affrontare e contribuire alla discussione che stiamo sviluppando non possiamo non sottolineare gli interrogativi che molti di noi si sono posti alla vigilia di questo dibattito, soprattutto in relazione al contesto politico nel quale esso si cala. Alcuni titoli dei giornali di oggi sono emblematici; ve ne è uno in particolare: il finimondo. Noi discutiamo cioè della riforma della Costituzione quando la situazione politica è caratterizzata certamente non da quelle condizioni che, in genere, si ricercano per affrontare temi di questa importanza e portata. Nel nostro Gruppo ci siamo molto interrogati su questo. Tuttavia, abbiamo voluto cogliere e lanciare anche una sfida: avviare una discussione su questi temi nel momento che apparentemente può sembrare quello meno opportuno. Per questo, penso

che gli uni e gli altri, affrontando questi temi, hanno compiuto, perché di fatto si sono tradotti in una totale inconcludenza. mio avviso, la prima questione che dobbiamo sconfiggere è questa caricatura che vede il Parlamento diviso in una metà dove ci sono i cosiddetti riformisti riformatori e in un'altra metà dove sono seduti i conservatori. Questa è una caricatura del Parlamento e della discussione che, nel corso degli anni che ci lasciamo alle spalle, abbiamo sviluppato

avendo in mente questo, credo che non andremmo da nessuna parte. Inoltre, nelle mozioni presentate c'è un punto che considero rilevante su tutti gli altri (non che i punti di merito che sono stati ricordati non valgano, ma su questi avremo tempo di effettuare un

per giungere alla necessaria approvazione di un testo condiviso dalla più ampia maggioranza parlamentare. Io considero questo il punto politico cruciale della discussione che c'è tra di noi, perché, ovviamente, in teoria siamo tutti d'accordo su questo, ma poi, passando alla prassi concreta, se guardiamo al passato non siamo molto incoraggiati. In realtà infatti, nell'affermare questo principio, dobbiamo anche essere consapevoli di una disponibilità non solo ad ascoltarci reciprocamente, perché questo lo facciamo normalmente in tante fondazioni, tanti centri studi e seminari nei quali ci ascoltiamo reciprocamente. Il punto è che dobbiamo avere la disponibilità politica a rinunciare a qualcosa a cui siamo affezionati, gli uni e gli altri, per giungere a un punto di sintesi. Vorrei quindi citare due punti su cui abbiamo discusso in passato e discutiamo ancora oggi:

riformare la giurisdizione e il suo modo di funzionare. Penso che tutte queste cose si reggano insieme. Il punto politico è capire quali sono i principi attorno ai quali pensiamo

Vorrei concludere questa riflessione dicendo che una repubblica presidenziale non è meno democratica di una parlamentare (potrei fare tanti esempi nel mondo); non è quindi su questo terreno che dobbiamo aprire il confronto tra di noi. Chi sceglie una forma piuttosto che l'altra lo fa perché dietro c'è una cultura, una storia, un assetto dei poteri, c'è un Paese formato in un certo modo. Penso che il senatore Nania abbia fatto bene a ricordare lo spirito che ha animato la Bicamerale, che ha affrontato questo tema e ha trovato un punto di sintesi; ad esempio, se noi riuscissimo a riesaminarlo, anche aggiornandolo, potremmo scoprire che si possono affrontare i temi della forma di Governo,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, è da molti decenni che stiamo dibattendo su questo tema, e potremmo risalire addirittura fino ai tempi della Commissione Bozzi. Ci auguriamo che questa sia una fase di decisione.

Poi il *referendum* non confermò quella riforma, quindi siamo sostanzialmente sempre al punto di partenza. La sinistra in altre legislature ha approvato parziali modifiche della Costituzione con un piccolo scarto di voti, peraltro con esiti che molti criticano, penso all'articolo 117 e ad alcune confusioni sorte nel rapporto tra Stato e Regioni, tant'è che molti si sono pentiti di aver voluto quella riforma. La bozza Violante di cui tanto si parla è comunque a nostro avviso un testo parziale, sostenuto oggi dalle attuali minoranze, che non possono pensare di imporre i contenuti di una riforma; altra cosa, giusta e ragionevole, è sviluppare un ampio confronto, che possa far emergere soluzioni condivise, visto che poi, a fasi alterne, una riforma più ampia ed organica della Costituzione, vuol dire che la mancata condivisione probabilmente è motivo non secondario del fallimento di un ampio disegno riformatore. Riteniamo, ad esempio, che l'istanza, la scelta, la vocazione presidenzialista sia importante. Sappiamo che non tutti convengono su questo aspetto, ma riteniamo che la democrazia diretta e il rafforzamento dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla scelta del Governo siano fondamentali. la Costituzione vigente in questo campo è in ritardo vistoso, perché la Costituzione materiale - quella che i cittadini pensano sia già in funzione - contempla già un'elezione diretta dei vertici di Governo. È inutile che mi dilunghi nel ricordare come le schede elettorali riportino vistosamente, a destra o a sinistra, i nomi dei leader dei candidati a Capo del Governo o come, pur permanendo una democrazia di tipo parlamentare, sarebbe inimmaginabile che un Presidente della Repubblica affidasse l'incarico di formare un Governo a persona diversa dal leader indicato dalla coalizione vincente (e difatti è sempre stata rispettata questa riforma sostanziale della Costituzione). Il presidenzialismo, quindi, è per noi anche garanzia di una democrazia matura, di un bipolarismo avanzato, che non deve essere archiviato, come temeva Panebianco giorni fa in un articolo sul «Corriere della Sera», ma un bipolarismo che deve essere consolidato come forma vincente e utile di democrazia governante dell'alternanza e anche della chiarezza nel confronto dei programmi politici. Le riforme quindi noi le vogliamo con convinzione, nel confronto e, se sarà possibile, anche nella condivisione delle scelte, come consolidamento di una democrazia più moderna e bipolare, basata su una volontà effettiva dei cittadini, al di là di alcuni bizantinismi dei riti parlamentari, che rispettiamo e che consideriamo fondamentali, che tuttavia richiedono anche questi una riforma. Non centrano le riforme costituzionali:

Abbiamo stilato un'agenda. Le mozioni che abbiamo scritto, lo sappiamo tutti, sono più un richiamo agli argomenti: non si possono sviluppare in questa fase le decisioni, che poi sono o saranno contenute nei disegni di legge presentati e in quelli

che riguarda il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, il tipo di funzioni dei magistrati, nel rispetto dell'autonomia della magistratura, evitando che si assista a terze Camere, che spesso si sovrappongono al Parlamento,

delle istituzioni parlamentari. Quindi, a nostro avviso, anche i temi della giustizia fanno ovviamente parte di questo indice di riforme e ci auguriamo che vi sia meno ritrosia nel confrontarsi. Il Popolo della Libertà, colleghi, è certamente convinto che uno dei punti fondamentali del suo programma, uno dei motivi della sua stessa nascita, origine e ragione di esistenza risieda in un processo di modernizzazione delle nostre istituzioni. Le riforme costituzionali sono nel DNA di una grande formazione politica riformista, che raccoglie varie esperienze e varie istanze e che, in questa legislatura, vuole arrivare a conclusioni reali. Gli altri colleghi del nostro Gruppo su altre tematiche nei loro interventi e il senatore Quagliariello, nella dichiarazione di voto finale, ribadirà queste e altre indicazioni. Noi cercheremo certamente il confronto, per le ragioni che ho voluto prima illustrare e richiamare. Se dalla Commissione bicamerale D'Alema fino ad altre fasi non si è mai arrivati a una conclusione, ciò vuol dire che, evidentemente, il confronto e la condivisione delle scelte possono essere un forte sostegno. Comunque, noi non consideriamo il confronto come un diritto di veto, perché riteniamo che le regole riguardino tutti: la maggioranza e, a maggior ragione, chi, alternativamente, si trova in minoranza nel Parlamento. Noi invitiamo soprattutto la sinistra a guardare con più coraggio a quegli obiettivi, anche presidenzialisti o di democrazia diretta, che anche oggi ho sentito da molti criticare ma che sono, invece, già presenti nel vissuto quotidiano del Paese. Non vogliamo decidere da soli, vogliamo confrontarci con tutti, ma rivendichiamo, comunque, il diritto-dovere di decidere in questa legislatura, visto che da decenni invochiamo riforme che poi non prendono corpo. Io mi auguro che anche questo dibattito ci impegni ad un confronto estenuante. Abbiamo già verificato, sul federalismo fiscale e su materie delicate che hanno un collegamento evidente con una diversa organizzazione della Repubblica, come sia stato possibile trovare occasioni di confronto e di convergenza. Noi le auspichiamo, non le escludiamo,

pensano sia già scritta nelle norme. Non aspettiamo ulteriormente per colmare questo distacco tra la Costituzione formale e quella materiale che gli italiani interpretano e sostengono con il loro voto.

Signora Presidente, prima di esprimere il parere, intendo anche dare un mio contributo alla discussione che si sta svolgendo oggi.

io segnalerei queste due iniziative, che io chiamo «le incompiute»: la riforma portata avanti dal sottoscritto nel 2006 (incompiuta perché non fu poi approvata dal *referendum* confermativo) e la riforma del 2001.

al di là delle modifiche al Titolo V, quelle postazioni che consentono al Governo di poter governare e al Parlamento di poter controllare e indirizzare l'Esecutivo.

il ricorso al voto di fiducia con i maxiemendamenti e l'opposizione viene accusata di sapere fare solo ostruzionismo. Ciò proprio perché forse, più che di poteri dell'Esecutivo e del Parlamento, sarebbe meglio parlare di poteri di veto incrociato e non di veri poteri.

Credo che questo sia il primo dei riconoscimenti, da una parte e dall'altra, del fatto che abbiamo sbagliato nel seguire questa strada. il dibattito che stiamo facendo quest'oggi, ma vorrei che non si fermasse all'aspetto formale e che si potesse riempire di qualche contenuto,

Credo che sarebbe il caso di verificare - anche al momento delle dichiarazioni di voto - se non ci sia la possibilità di addivenire a un' unica mozione.

non è il caso di pensare a un'Assemblea costituente, visto che non siamo a ridosso della conclusione di un conflitto. Lo strumento delle Bicamerali forse porta davvero male, perché gli argomenti trattati poi finiscono in niente. A me era venuta in mente in passato un'ipotesi, che propongo non come impegno del Governo, ma come argomento di riflessione: e se si utilizzasse, ad esempio, una Convenzione costituente, ovvero

gli articoli che, in modo condiviso, intendiamo modificare e per provare a scrivere un testo che possa avere poi un passaggio parlamentare in forma magari più semplice rispetto all'esame ordinario.

i numeri relativi ai tempi necessari per l'approvazione media di una legge ordinaria e il numero delle leggi ordinarie che vengono approvate rispetto alla decretazione d'urgenza, ci si rende conto che

che quelle riforme dei Regolamenti parlamentari - in tante occasioni discusse e tentate, e poi mai realizzate - debbano essere invece costituzionalizzate: se c'è e deve esserci - come io ritengo - una corsia preferenziale per l'esame di argomenti indicati dal Governo, questa deve esistere indipendentemente dalla volontà o meno di una maggioranza che, in

alle corsie riservate e preferenziali, non solo per l'esame delle iniziative parlamentari dell'opposizione, ma anche di quelle di maggioranza; oggi infatti il Parlamento soffre da una parte e dall'altra l'unica attività legislativa, o quasi, è quella della decretazione d'urgenza. Riconosciamo allora al Parlamento quella possibilità, da una parte e dall'altra. Un altro aspetto che ritengo rilevante

«e della necessità di approvare una conseguente legge elettorale che contempli il principio di rappresentanza». parere favorevole sulle mozioni nn.

Signor Presidente, colleghi, credo ognuno di noi, e in modo particolare il sottoscritto, se ne andrà deluso da questo dibattito. È una sconfitta per il Parlamento. Dovevamo a tutti i costi puntare ad un documento comune. Era stato proposto da qualcuno di noi

siamo convinti tutti - destra, sinistra, centro - che non è più possibile fare le riforme a maggioranza. Non è che le rifiuta un partito politico: le rifiuta la comunità nazionale; ce lo ha dimostrato in tanti modi e ce lo dimostra tutti i giorni. Le regole in un Paese civile e democratico devono essere regole condivise da tutti.

Riproporre, invece, un Esecutivo più forte, che abbia la possibilità di decisioni più veloci per rispondere alle esigenze della società, credo sia giusto. Ancora una volta, mi è sembrato di vedere troppi tatticismi attorno a questa materia. Credo però sia giunto il momento in cui ognuno di noi è chiamato a grandi responsabilità. Ecco perché ci vogliono posizioni concrete. Lei, signor Ministro, diceva quale poteva essere il sistema per modificare la Costituzione. Perché no? Quello che lei ha proposto - convenzione costituente - o addirittura,

(perché in Italia sono anche troppe le forme di governo locale) che portino all'aggregazione di interessi, magari territoriali. Questa è la sfida. Siamo pronti tutti; ma, purtroppo, stasera ne usciamo con posizioni totalmente diverse.

l'onestà intellettuale con la quale ha posto alcune questioni, non da ultimo quella relativa al ruolo del Parlamento nel suo rapporto con un Esecutivo più forte. Certamente ci avrebbe fatto piacere ascoltare dalla sua voce la giusta rivendicazione di un taglio non solo del cosiddetto sistema dei costi della politica, ma anche, ad esempio, delle Province che, così come sono, non funzionano e non servono a niente. a niente. Perché l'Unione di Centro ha condiviso con il Partito Democratico una mozione che impropriamente ed erroneamente è stata definita minimalista? Proprio per e nel tentativo di riprendere il cammino delle riforme e di riprendere il bandolo della matassa, partendo da un punto certo: il fallimento di tutte quelle ipotesi riformatrici che sono state portate avanti a colpi di maggioranza. La prima questione centrale che viene posta all'attenzione del Senato è proprio fino a quando le riforme costituzionali ed istituzionali si faranno con il vincolo di maggioranza, quelle riforme sono destinate a durare lo spazio di un mattino. Ciò è avvenuto

Quella riforma ha fatto crescere in maniera disordinata il sistema istituzionale, il quadro dei rapporti e il sistema delle competenze fra Stato, Regioni ed autonomie, a tal punto che oggi il Governo centrale, per condurre e guidare alcuni processi fondamentali in materia di risanamento economico e finanziario, deve fare violenza sulle Regioni, che hanno mostrato limiti enormi nella gestione della spesa sanitaria e di settori fondamentali relativi ai servizi a vantaggio dei cittadini. Analogo fallimento Analogo fallimento si è registrato con la riforma del centrodestra. Mi rivolgo senza polemica ai sacerdoti della sovranità popolare. caso è successo un fatto che non può essere taciuto, altrimenti sviliamo il senso e ci trinceriamo dietro l'ipocrisia di questo dibattito. Quella fu la prima volta che una riforma ampia della Costituzione fu sottoposta al voto popolare e la maggioranza assoluta dei cittadini italiani, partecipando al *referendum*, bocciò quella proposta. Poiché tutti noi siamo legati al principio del rispetto della sovranità popolare, quello è un altro punto fermo nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali. vuole segnalare la nostra mozione sul piano del perimetro e del metodo di confronto su un tema estremamente delicato. Noi abbiamo proposto di partire dalla bozza Violante non perché questa sia la panacea di tutti i mali,

favorevole della maggioranza parlamentare di allora, di cui il mio partito non faceva parte, e un voto di astensione dei quattro partiti all'epoca all'opposizione: Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC e Lega.

di impegnare il Governo sul tema delle riforme sia impropria. Noi, proprio per un approccio non ipocrita al tema delle riforme, abbiamo coinvolto nel dibattito parlamentare il Governo, perché è che, per conto della maggioranza, sta guidando il processo riformatore all'interno delle nostre istituzioni. Poiché il futuro delle riforme, così come lo è stato per il federalismo fiscale, al destino di questa maggioranza, sarebbe ipocrita pensare che il Governo assuma una posizione terza rispetto a un dibattito che, proprio perché oggi ha sperimentato tutte le strade possibili nella democrazia del maggioritario (tutte fallimentari), ha bisogno di ricondurre tali strade all'essenzialità, alla serietà e alla possibilità di una condivisione di alcuni aspetti fondamentali. A tale riguardo, perché abbiamo segnalato solo tre questioni nella mozione?

del Senato federale è un'ipotesi sulla quale abbiamo sempre avuto grandi perplessità. Tuttavia, è evidente che, se dobbiamo trovare le ragioni che uniscono e non quelle che dividono, dobbiamo sfrondare il dibattito e riportarlo, intanto, a quel minimo comune denominatore che serve ad avviare in maniera chiara e precisa il tema delle riforme costituzionali. La riduzione del numero dei parlamentari, l'idea di un Senato federale o delle Regioni, comunque ancorato al territorio e al sistema delle competenze, così come è stato scritto nell'articolo 117 della Costituzione, nella riforma del Titolo V (che comunque andrebbe migliorato), sono patrimonio condiviso della maggioranza e delle opposizioni. Anche il tema del superamento del bicameralismo perfetto è patrimonio condiviso; peraltro, sia nella cosiddetta bozza Violante che nella riforma del centrodestra del 2006, la questione è stata affrontata con grande serietà anche sotto il profilo tecnico, e credo che sia comunque un buon punto di partenza per arrivare ad alcune conclusioni. Se non si hanno pregiudizi e riserve.

darebbe uno stimolo in più. Noi siamo aperti, signor Ministro: questo confronto lo vogliamo portare avanti senza riserve e pregiudizi, a 360 gradi. Per questa ragione pensiamo che anche il tema della giustizia e il rapporto tra politica e magistratura,

vale per il tema del premierato forte con un Parlamento forte, con organi di garanzia costituzionali o di rilievo costituzionale degni di questo nome. Pensiamo al dibattito che vi è stato

costituzionali, io credo che il senso sia quello di dare risposte in termini di maggiore efficienza e trasparenza ai cittadini che ne hanno bisogno. Per questo spero e mi auguro, signor Presidente, che si possa arrivare ad un unico testo, così come il ministro Calderoli ha proposto.

il dibattito culturale e politico degli anni più recenti è stato spesso dominato dall'illusione che le riforme istituzionali potessero essere la chiave universale, lo strumento necessario e sufficiente per risolvere gran parte dei problemi dei Paese. Occorre invece essere consapevoli anche dei limiti delle riforme istituzionali. Esse non sono la panacea di tutti i mali della nostra democrazia. Non possono sostituire l'iniziativa delle forze politiche, la loro capacità di riformare se stesse e di ristrutturare nel contempo l'assetto del sistema politico nel suo complesso: i processi politici, senza escludere quelli di moralizzazione, possono produrre effetti anche più rilevanti di quelli prodotti dal cambiamento delle sole regole e degli assetti istituzionali. Del resto, nell'ambito di un dibattito parlamentare sulle riforme costituzionali, occorre doverosamente premettere che, purtroppo, la vita quotidiana dei cittadini italiani non risente - almeno nel brevissimo periodo, caratterizzato dall'aumento della disoccupazione e dall'aumento dell'inflazione - del mutamento della forma di Governo o della revisione del bicameralismo perfetto. Detto in termini più espliciti, a pancia vuota, delle riforme non interessa molto alla gran parte del Paese. Il «giorno per giorno» dei cittadini risente invece, moltissimo, dei livelli di efficienza dei servizi pubblici come la giustizia, il lavoro, la sanità, la scuola, la ricerca, i trasporti, oltre che del grado di vivibilità delle nostre città. Questi si possono raggiungere con buone leggi ordinarie, senza stravolgere i canoni costituzionali. Le risposte che il sistema politico nel suo complesso ha il dovere di fornire ai cittadini italiani proprio nella Costituzione repubblicana e nei suoi insuperabili principi di giustizia, uguaglianza ed equità, che possono tradursi in leggi e provvedimenti concreti a partire dalla riforma della legge elettorale per arrivare a quella per superare i conflitti di interesse, da quello del Presidente del Consiglio a quello dell'ultimo consigliere di circoscrizione. Dobbiamo dare atto il presidente Colombo lo ha ribadito - alla nostra Costituzione di avere conservato fino ad oggi il suo straordinario valore, preservando, attraverso le trasformazioni realizzatesi in oltre sei decenni, la sua tenuta con riconosciute, prudenti elasticità e attitudini a comprendere fenomeni non prevedibili dai costituenti. Nella consapevolezza che la prima parte della Costituzione, contenente i principi fondamentali, non è indipendente dalla seconda, che contiene le norme organizzative che servono a farli valere o che, comunque, ne condizionano l'attuazione, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che qualche aspetto della Parte II si possa certamente discutere e rivedere, nel rispetto di quelli che riteniamo essere i valori supremi sottesi alla nostra Costituzione. La scelta di interventi limitati ad alcune questioni, anche se di notevole portata, apparirebbe oltretutto conforme conforme alla corretta lettura dell'articolo 138 della Costituzione, così come sottolineato da dottrina attenta e condivisibile, che impone revisioni costituzionali circoscritte e dotate, comunque, di una matrice omogenea e tra loro unitaria. Ecco perché riteniamo che gli interventi dovrebbero concentrarsi su alcune significative questioni, come la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, la limitazione dei mandati dei parlamentari, la modifica della composizione e delle funzioni del Senato della Repubblica e la conseguente modificazione del procedimento della formazione delle leggi, l'incandidabilità dei condannati, un insopprimibile principio di equilibrio tra i poteri dello Stato. La mozione del Gruppo dell'Italia dei Valori non formula un impegno all'Esecutivo: i colleghi Pardi e Li Gotti lo hanno ribadito. Noi riteniamo fondamentale che il Governo non debba incoraggiare nessun *iter* legislativo perché questo connota i principi della nostra democrazia parlamentare.

e non possiamo accettare un'idea di revisione della Costituzione che voglia, da un lato, rafforzare i poteri dell'Esecutivo e, dall'altro, rivedere norme di «rango costituzionale che sovrintendono al funzionamento del nostro sistema giudiziario». no a maggiori poteri all'Esecutivo. Anche le recenti riforme costituzionali approvate in Francia e proposte in Gran Bretagna esprimono l'esigenza non di ribaltare, quanto piuttosto di riequilibrare il rapporto tra Esecutivo e Legislativo là dove sbilanciato a causa della eccessiva concentrazione di poteri del primo a scapito del secondo. L'Italia dei Valori ritiene che non ci sia assolutamente bisogno di un rafforzamento del potere dell'Esecutivo, perché ormai questo, per come ne degradata l'interpretazione, va occupando qualsiasi spazio. Lo strumento della decretazione d'urgenza, accompagnato dall'uso abnorme della questione di fiducia, spesso su maxiemendamenti che riscrivono i testi legislativi sottraendo al Parlamento ogni possibilità di ulteriore approfondimento e modifica, ci dice che non abbiamo nessuna necessità di ampliare i poteri dell'Esecutivo. no alla revisione delle norme costituzionali in materia di giustizia. È inaccettabile per l'Italia dei Valori e per il Paese il ritorno alla vecchia immunità parlamentare, privilegio castale dotato oggi, e non allora, di totale irragionevolezza e di mancanza di buonsenso. Inaccettabile per l'Italia dei Valori e per il Paese è la separazione delle carriere dei magistrati. Inaccettabile per noi e per il Paese è che la polizia giudiziaria venga di fatto sottratta al controllo della procura e indirettamente ricondotta, tramite la catena gerarchica, al controllo dell'Esecutivo. Inaccettabile è, in definitiva, che i giudici e l'ordinamento giudiziario vengano intesi come opposizione politica da distruggere ed abbattere. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'importante tema della riforme costituzionali non può diventare un ossimoro insensato utilizzabile dalle forze politiche per giustificare solo a parole atteggiamenti o vaghe ideologie. Esso deve invece rappresentare l'occasione attraverso cui le forze politiche prendano coscienza del Paese, delle sue realtà, delle sue difficoltà, specie in questi momenti di spaventosa e perdurante crisi. Il Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori vuole esserci. Vuole essere, cioè, forza propulsiva per migliorare l'efficienza istituzionale del Paese, ma senza picconare nulla. Collega Astore, sei stato un anno e mezzo nei banchi dell'opposizione: la tua esigenza di rafforzare l'Esecutivo mi fa intendere che tu non abbia capito una lezione che abbiamo cercato di studiare insieme per un anno e mezzo. Per recuperare il senso, oggi sempre più sbiadito, di una democrazia rappresentativa, oggi abbiamo bisogno di discutere, ma non di stravolgere. Concludo, signor Presidente.

alcune mozioni che vedranno il nostro voto contrario, perché - ripeto - non abbiamo bisogno di stravolgimenti della nostra Carta costituzionale, il cui insegnamento è marchiato nelle nostre coscienze e intendiamo tramandarlo anche ai nostri figli. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voglio ringraziare innanzitutto i colleghi Capogruppo della maggioranza - il senatore Gasparri, il vice capogruppo del PdL senatore Quagliariello e il senatore Pistorio - per il lavoro che hanno svolto insieme a noi nella fase preparatoria di questa mozione. Voglio ringraziare anche i Capigruppo dell'opposizione - il senatore D'Alia ed in particolar modo la senatrice Finocchiaro - per aver richiesto la calendarizzazione di queste mozioni e per aver contribuito a questo costruttivo confronto parlamentare. Oggi, con l'approvazione di queste mozioni, abbiamo fatto un passo sicuramente importante verso quel cambiamento richiesto dai cittadini, a nostro avviso ancora più rilevante perché fatto in un clima politico di forte contrapposizione. L'importante - e come Lega lo abbiamo sempre detto - è evitare che lo scontro politico che è in atto tra maggioranza e opposizione interferisca e blocchi la strada delle riforme costituzionali. Su questi temi, per quanto ci riguarda, è giusto e doveroso, almeno in Parlamento, fare tutti un passo indietro per avviare un confronto serio e costruttivo in grado di portarci ad un testo di riforma condiviso per cambiare insieme questo Paese. Ci si può scontrare su tutto, ma non sulle riforme costituzionali. Dico questo perché parto da una considerazione a mio avviso molto importante: in passato la mancata intesa tra maggioranza ed opposizione - è stato ricordato prima anche dal ministro Calderoli e da altri interventi - ha fatto naufragare tutte le iniziative di riforma affrontate in Parlamento. Tutte. Anni di lavoro, di discussioni, di dibattiti nelle Aule parlamentari, nelle Commissioni, supportati da indagini conoscitive, da comitati di esperti, alla fine hanno prodotto solo un fiume interminabile di parole, ma mai nessun risultato. Anche le varie Commissioni bicamerali hanno fallito il loro obiettivo; ricordo la più famosa, quella guidata dall'allora presidente D'Alema. Stessa sorte per le riforme votate a colpi di maggioranza, come quella della modifica del Titolo V della Costituzione, voluta dal centrosinistra, che, a detta di tutti, si può definire incompleta e lacunosa. O quella sulla *devolution*, votata dal centrodestra e bloccata poi dal *referendum* confermativo. Dopo vent'anni di discussione i risultati sono pari allo zero: questa è la realtà. È dunque evidente che, se si vuole raggiungere l'obiettivo non solo a parole ma anche nei fatti, l'unica strada da percorrere è quella delle riforme condivise. Basta dunque con gli scontri inutili; basta con le riforme a colpi di maggioranza. Abbiamo sicuramente un vantaggio nei confronti delle esperienze negative del passato: su molti temi oggi la pensiamo allo stesso modo. Penso alla fine del bicameralismo perfetto (dunque all'istituzione di una Camera delle Regioni o di un Senato federale), alla riduzione del numero dei parlamentari, a una forma di governo più moderna, ferme restando le prerogative di controllo del Parlamento. Fino a pochi anni fa, solo la Lega portava avanti queste proposte. Oggi, almeno a parole, tutti si dicono convinti che queste riforme sono necessarie al Paese, che non sono più rimandabili, che sono l'unica via d'uscita, anche perché - diciamolo chiaramente - i primi a chiederle con forza e determinazione sono i cittadini. È dal popolo che è partita questa spinta riformatrice. *(Applausi le chiedono gli elettori del centrodestra e del centrosinistra, ma non solo: le chiedono con forza tutto il Nord unito e anche le Regioni del Mezzogiorno. Ormai è tutto il Paese che le pretende: questa è la realtà dei fatti. Allora, se siamo convinti di questo, mettiamoci a lavorare. Abbiamo tutto il tempo per discutere ed approvare le riforme: davanti a noi abbiamo tre anni e mezzo di legislatura, ma se troviamo un accordo le si possono fare in molto meno tempo, anche perché di tempo, come Paese, ne abbiamo perso fin troppo. Basti pensare al diverso cammino delle riforme realizzato con successo nelle altre democrazie occidentali. In tutti gli Stati europei si registrano fenomeni di amplissima regionalizzazione accomunati dalla medesima finalità istituzionale: la valorizzazione delle autonomie territoriali. Ai tradizionali ordinamenti federali (mi riferisco alla Svizzera, alla Germania e all'Austria) si sono affiancati nel tempo fenomeni federativi come quelli del Belgio e della Spagna, per citarne alcuni, che sono emblematici, per il nostro dibattito interno, di un diverso approccio al federalismo, non secondo il tradizionale patto federativo fra Stati membri preesistenti, tipico dell'esperienza statunitense e di quella tedesca, bensì mediante un processo di riforma dello Stato centrale in uno sempre più federale. Questi passaggi fondamentali, che vanno a modernizzare la struttura dello Stato per renderlo più efficiente e in grado di ridurre la spesa pubblica e gli sprechi, in Europa tutti li hanno già superati da anni, in molti casi da decenni.

Abbiamo anche la fortuna di avere un Governo unito e deciso sulle riforme da realizzare, perché le ha inserite nel proprio programma elettorale. Saranno il ministro Bossi con il ministro Calderoli a seguirle passo passo, e questa è sicuramente un'ulteriore garanzia. Lo dico perché i ministri Bossi e Calderoli hanno dimostrato nella riforma del federalismo fiscale la massima attenzione al lavoro del Parlamento partecipando a tutte le sedute di Commissione senza delegare nessuno, ascoltando tutti, soprattutto le opposizioni. è giusto ricordarlo - ci ha permesso di approvare una riforma importante come quella federalismo fiscale al Senato senza voti contrari, cosa mai avvenuta in passato. passato. Diciamolo chiaramente: se c'è davvero la volontà di fare le riforme non ci sono scuse. Se invece si desidera sfruttare il tema delle riforme costituzionali per trovare pretesti per alimentare lo scontro politico in questo Paese, allora è un altro discorso. Chi lo farà se ne assumerà tutta la responsabilità; dico solo che la Lega non parteciperà a questo gioco politico. sono temi troppo importanti per essere strumentalizzati. Siamo convinti di essere di fronte a un'occasione storica, quella di cambiare il Paese, e nessuno ci farà cambiare idea. Le polemiche, per quanto ci riguarda, sono solo tempo perso. Lo abbiamo dimostrato in questi mesi non partecipando al dibattito politico che si è concentrato sui *gossip*, sulle veline e sugli scandali. Non siamo intervenuti neanche quando erano i rappresentanti dell'opposizione a esserne colpiti, e penso - uno su tutti - al caso Marrazzo. Non ci interessano queste polemiche, siamo convinti che i cittadini si meritino altro. E voglio essere ancora più chiaro, e mi rivolgo soprattutto ai tanti giornalisti che cercano in tutti i modi di avvelenare, se possibile ancora di più, il clima politico in questo Paese, cercando di creare contrapposizioni tra noi e gli altri Gruppi parlamentari. Noi non siamo al Governo e in Parlamento per litigare, né con la maggioranza, né con le opposizioni: noi siamo in Parlamento per cambiare finalmente questo Paese e per fare le riforme. Non ci interessa altro. Detto questo, che è importante perché alle polemiche non ci siamo stati in quanto siamo convinti di quello che stiamo facendo al Senato e in Parlamento, ci auguriamo che le mozioni di oggi possano segnare l'avvio di una nuova fase, detto, sul dialogo e sul confronto, senza più i veti incrociati del passato, senza contrapposizioni inutili e sterili. Riusciremo così a centrare questo obiettivo. Faremo un servizio al Paese e ai cittadini onesti che pagano le tasse e che ci chiedono come politica risposte concrete. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Calderoli, consideriamo l'occasione di oggi una buona occasione, politica innanzi tutto, utile per l'Italia. È un'occasione che abbiamo cercato, assumendone l'iniziativa ed anche la responsabilità, perché vediamo con gli stessi occhi con i quali gli italiani guardano alla scena pubblica ed alla scena istituzionale quale sia la rappresentazione che ogni giorno si manda in scena: quella di un conflitto perenne ed improduttivo, dove a vincere è solo la tentazione di far prevalere la forza, anche - direi soprattutto - su un terreno, quello delle riforme istituzionali, che dovrebbe essere messo in salvo, tenuto al riparo dalla contingenza dello scontro. Scontro che è tutto legittimo, naturalmente, tra opzioni diverse sulle singole questioni e sulla stessa gerarchia tra le priorità da affrontare. l'ispirazione di oggi, lo voglio dire con chiarezza, non è una riedizione di quel dialogo di cui si è brevemente favoleggiato all'inizio della legislatura: una parola che ci è rotolata in bocca come una caramella appiccicosa e dolciastra. Né è tantomeno, lo voglio dire con ogni chiarezza, uno scambio: non c'è nessuno scambio! Noi siamo contrari al processo breve, lo stiamo mostrando con le armi tipiche dell'opposizione, con il nostro ostruzionismo, e lo mostreremo con i nostri emendamenti, ed ancora una volta cercheremo di risolvere la questione (pretesa) della lunghezza dei processi con riforme di sistema che non la danneggino, ma che rendano davvero più celere la giustizia. Noi siamo però anche quelli che non conoscono altro diritto di difesa che quello che si esercita nel processo e che però crediamo nei valori del garantismo. Siamo quelli che non cercano le scorciatoie giudiziarie e che sanno distinguere tra il livello della responsabilità politica e il livello della responsabilità penale. Mi permetto di dire, con la mia modestissima esperienza, che chi ha provato ad essere giudice, sforzandosi di esserlo al meglio delle proprie forze, sa davvero distinguere, ancora e meglio, colleghi, tra il profilo della responsabilità penale ed il profilo della responsabilità politica, e che questo non toglie niente, nessuna forza alla durezza del giudizio politico. Noi siamo questo. Contrastiamo le leggi singolari e chiediamo riforme di sistema. In questo esponiamo noi stessi e la nostra responsabilità di maggiore partito dell'opposizione. Ci opponiamo all'indebolimento dell'ordinamento, frammentato da troppi provvedimenti contingenti (magari adottati per interessi particolari) e offriamo la nostra forza per rendere forte ed efficace il sistema. Io non vedo contraddizione in questo. Semmai, colleghi, vedo coraggio, perché ci vuole coraggio a non essere, dall'opposizione, forza di blocco e perché non è la conservazione il nostro riparo Quindi, riforma di sistema, quindi un luogo perché questa riforma possa farsi. È necessario, e ne hanno parlato in tanti. ne ha parlato il ministro Calderoli, che io ringrazio per l'intervento di merito e anche, mi lasci usare questo termine, per che ha fatto oggi, e ne hanno parlato molti colleghi. Le Commissioni bicamerali, che sono state ricordate negli interventi precedenti, datano ormai a qualche decennio. due riforme costituzionali, una operata dal centrosinistra e l'altra dal centrodestra, sia pure per ragioni diverse, sono state approvate con strettissima maggioranza. É stato così. Oggi noi ci troviamo nella necessità - io credo - di sconfiggere quel rischio che il presidente Napolitano così spesso e e con tanta serietà e autorevolezza ci rappresenta: il rischio di una reciproca delegittimazione continua, il rischio di un collasso istituzionale. Allora, mettiamoci alla prova, opposizione e maggioranza. Io ritengo, nonostante il fatto che non si sia arrivati a una mozione unica (rispetto alla quale vi era la nostra disponibilità, ovviamente nella differenza delle posizioni),

affinché le riforme costituzionali in questo Paese si facciano, da questo momento in poi, a larga maggioranza. Questa non è l'ovvietà, in questo tempo della politica, ed invece è giusto che così sia. Lasciatemi anche dire, di fronte alle obiezioni dei colleghi radicali e di altri colleghi, che io non solo comprendo ma assumo pienamente nel loro valore, che la stessa forma scelta della mozione non è casuale, ma nasce dal contesto. intenzione polemica, ma troppe volte ci siamo sentiti dire dal Capo del Governo che le riforme si sarebbero fatte a maggioranza e che la maggioranza bastava a sé sola per riformare la Costituzione. Il coinvolgimento pieno del Governo tiene conto di questo e anche del fatto che quando questo impegno viene assunto è un impegno sul quale abbiamo ricevuto anche una compiuta espressione del ministro Calderoli.

partecipazione che lei ha visto, sperimentato e assecondato durante la discussione del provvedimento sul federalismo fiscale. C'è un punto di differenza, il primo e forse più significativo, tra la nostra mozione e quella presentata dai colleghi della maggioranza. Esso riguarda la riforma elettorale.

che la questione della riforma elettorale non attiene soltanto alle conseguenze di un quadro che potrebbe mutare - l'abolizione del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari - ma attiene a un'esigenza che io sento più profonda, e lo dico anche ai colleghi della Lega l'esigenza di ripristinare in questo Paese quel principio essenziale di ogni democrazia, di riannodare il filo della rappresentanza politica e di tornare a parlare, colleghi della Lega Nord, di una responsabilità degli eletti nei confronti dei loro elettori e non del segretario di partito che li ha messi in lista. Quindi, rivendico con questa parte della mozione, insieme ai colleghi firmatari, una pretesa democratica, ma non mi fermo a questo, perché vediamo un nesso stretto tra il ripristino del principio di rappresentanza e tanta parte delle questioni che attengono al ruolo e alla medesima funzionalità del Parlamento, alla sua efficacia, alla sua missione costituzionale. Certo, i colleghi hanno introdotto il tema dei Regolamenti parlamentari, di cui ha parlato il presidente Gasparri: siamo d'accordo e sosteniamo questa discussione, che anzi vorremo fosse più celere e produttiva, in tempi brevi, di un testo. Certo, ragioniamo ancora del superamento del bicameralismo paritario, anche in ragione degli impegni che ricordava il presidente Bricolo e che abbiamo assunto con l'approvazione del federalismo fiscale e ragioniamo di rafforzamento del Parlamento insieme a un rafforzamento dell'Esecutivo. Ma perché voglio attirare l'attenzione dei colleghi su questo punto, per spiegare la cura che abbiamo nel menzionare tale questione? Lo faccio non con un'idea di parte, ma cercando di ampliare l'orizzonte e lo sguardo della nostra riflessione. Vedo infatti il rischio che oggi il Parlamento resti stretto tra due

di lasciare non solo integro, ma forte, rappresentativo e incidente il ruolo del Parlamento, secondo la missione costituzionale che è iscritta nelle regole tra di noi condivise. C'è poi un punto che riguarda l'ordinamento giurisdizionale. Noi ovviamente insistiamo perché non si scompagini in nessun modo l'equilibrio tra i poteri, quell'impianto resti preservato e l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario siano in ogni modo garantiti.

che in realtà abbiamo già affrontato e che il Parlamento ha già discusso quando abbiamo operato la riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal ministro Castelli, che solo in parte è stata poi modificata nella successiva legislatura, preservandone peraltro i capisaldi.

preferito: era il traguardo e l'obbiettivo che mi prefiggevo, però, sin dall'inizio, già in partenza, ho avvertito prioritariamente la necessità di accostarmi a questi temi e al dibattito di oggi

con la cura che si deve a un oggetto fragile, a una questione assai delicata, che appartiene e che può descrivere il futuro e le occasioni dell'Italia. Do atto alla maggioranza, nonostante non si sia arrivati ad un testo condiviso, di avere compreso e condiviso questa cura che poi si manifesterà nelle modalità di voto. Non siamo arrivati - e forse il tempo che seguirà questo intervento ci dirà qualcos'altro - ad un testo condiviso, ma io ho già misurato che abbiamo registrato sulla stessa lunghezza d'onda la cura e l'attenzione con cui ragioniamo. Ci sarà quindi una condizione di reciprocità nell'atteggiamento di voto che, proprio per questo, darà maggiore forza all'impegno comune dell'approvazione a larga maggioranza delle riforme costituzionali. Certo, oggi è solo un *incipit*, ma è già un inizio.

ma avremo rotto il blocco delle nostre contrapposizioni, che blocca l'Italia e la ferma. Sposteremo su un altro livello la discussione politica. Bisogna capire se ne ne saremo capaci fino in fondo. Qui sta la scommessa per noi e per voi, esattamente nello stesso modo. Possiamo restare impastoiati, lo dico ai colleghi della maggioranza, nelle mille trappole avvelenate dei mille veleni che hanno segnato questi anni, con 18 tappe, 18 provvedimenti singolari, oppure si possono affrontare i nodi di sistema e i temi delle riforme. Frammentare un sistema o contare sulla forza e l'autorità di un sistema che funziona e che insieme riscriviamo. peraltro che questo sia anche il compito di un grande partito riformista, come il Partito Democratico, e questo anche oggi abbiamo cercato qui di testimoniare. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, accetto l'invito alla cura. Questa è una prima occasione. Per non sprecarla è necessario dire poche cose e compiere un atto di buona volontà. E allora, per dire poche cose ma chiare, diremo innanzitutto che la Costituzione per noi non è un totem, non è un mito intangibile. È un grande accordo politico come tale datato ed emendabile. Ci è stata affidata in un momento storico particolare e molto difficile per il nostro Paese dai Padri costituenti, che hanno lasciato alle future generazioni il compito di definire tre capitoli che loro non erano riusciti a definire. Basta rileggersi il "testamento" di Meuccio Ruini, colui il quale più di ogni altro ha contribuito al compromesso della seconda parte:

ha fatto sì che, per scongiurare l'instaurazione di una sorta di regime assembleare, che pure è un rischio presente nell'equilibrio dei poteri della si realizzasse quella che Pietro Scoppola definì la Repubblica dei partiti, assurti di fatto al ruolo di fulcro del sistema istituzionale. Quei partiti erano qualcosa di più che istituzioni di fatto. Erano anche aggregati sociali. Si chiamavano anche partiti di integrazione sociale perché in quei partiti si viveva una parte della propria esistenza, si passava persino una parte del proprio tempo libero. Ora, quei partiti sono finiti, travolti non tanto e non solo dai grandi cambiamenti istituzionali, ma soprattutto dai grandi cambiamenti sociali, sociali, travolti dalla modernizzazione, che ha chiuso le sezioni di paese in cui una volta si giocava a carte. Dal 1994, e più decisamente dopo il 2008, il sistema politico italiano ha virato verso una democrazia degli elettori: una situazione sostanziale, suggellata dalla volontà dei cittadini, dalla ricerca di un contatto diretto tra gli elettori e la rappresentanza, che esiste e vive nei fatti, nei simboli, anche se non ha trovato ancora un sua codificazione istituzionale. Questa per noi è la sfida che ci troviamo di fronte: non si tratta di razionalizzare un sistema ormai superato, che ha avuto i suoi grandi meriti storici, ma di organizzare e di dare forma istituzionale ad un'evoluzione sociale, che si è prodotta naturalmente. Non si tratta, dal nostro punto di vista, di compiere strappi, ma di procedere consapevolmente lungo la strada della modernizzazione.

senza esclusione, un rapporto diretto tra il potere esecutivo e il corpo elettorale. Ed anche quando questo rapporto è sancito da un'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Capo del Governo, il ruolo fondamentale del Parlamento, dell'Assemblea legislativa, non è messo in discussione. Piuttosto, se si vuole che il Parlamento conservi la sua centralità e, anzi, tragga nuovo impulso dalle nuove regole, che mi auguro andremo a scrivere insieme, sarà importante non solo metter mano ai suoi meccanismi di funzionamento, ma anche individuare la strada migliore per superare il bicameralismo perfetto.

Gruppo* *PdL)*. Quando si è giunti ad immaginare un Senato estraneo al circuito della fiducia, ci si è posti lungo un sentiero impervio, con due sole alternative: dar vita ad un Senato subordinato all'altro ramo del Parlamento, o attribuire ad esso un «potere contrattuale» nei confronti dell'Esecutivo, giocato inevitabilmente sulla pelle del debito pubblico. Infine, se si vuole davvero intraprendere un cammino di riforma che modernizzi il nostro Paese e lo renda una democrazia "normale", non si può espellere il capitolo della giustizia. Apprezzo le aperture in tal senso contenute nell'intervento della presidente Finocchiaro. Infatti, se ci si richiama alla Costituzione e allo spirito che ne ha animato la stesura, non sono ammesse censure: si deve prendere atto che l'articolo 68, pensato dai Padri costituenti, serviva a introdurre nel sistema un elemento di equilibrio fra l'ordinamento giudiziario e la vita politica. Guardiamoci intorno senza paraocchi ideologici: vi sono soluzioni diverse, ma nessuna grande tradizione costituzionale omette di porsi il problema di questo equilibrio e di come evitare che poteri fondamentali dello Stato entrino in conflitto. Il problema, insomma, non è soltanto quello di garantire loro un seppur sacrosanto spazio di autonomia.

ma di preservare la sovranità del popolo. Non si tratta di svincolare il potere politico da un equilibrio di pesi e contrappesi, ma piuttosto di ricreare quei pesi e contrappesi che i Padri costituenti avevano non a caso immaginato. Soprattutto, non si tratta di una sola persona, ma della stabilità delle nostre istituzioni, dello sviluppo del nostro Paese, del futuro della nostra democrazia.

Non faremo mancare il nostro contributo per la riforma americana delle istituzioni, per il sistema elettorale anglosassone se, quando e dove tale dibattito ci sarà. Oggi faremo invece mancare il nostro sostegno a questo metodo, all'irritualità di questo dibattito. Il nostro voto contrario è per rafforzare la centralità del Parlamento, la dignità delle istituzioni svilite

Se c'è la volontà di cambiare la Costituzione, questo è il luogo. A noi senatrici e senatori spetta il compito di fare proposte politiche precise, non chiedendo al Governo di essere accompagnati per mano come bambini. È avvilente che lo chieda la maggioranza; è incomprensibile che però lo solleciti l'opposizione. nuova finestra"). Prima di procedere alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Vi sono tutti i presupposti perché dal Senato possa partire una fase costituente, come ci chiedono gli italiani. Lo abbiamo sempre sostenuto, così come abbiamo sempre sostenuto che sui testi, sulle idee e sulle proposte ci si poteva trovare assieme. Questa sera abbiamo dimostrato che questo percorso è possibile. Vi ringrazio.